L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. In data 15 dicembre 2021, il Primo Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ha inviato la seguente lettera: «Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ho l'onore di comunicarLe che in data odierna il Collegio previsto dal medesimo articolo 2, lettera *b*), ha eletto giudice della Corte costituzionale il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi.

Presidente, ho chiesto la parola per ricordare Marco, Roberto e Filippo, le tre persone che hanno perso la vita sotto una gru a Torino. Soltanto qualche mese fa ricordavamo Luana, impressionati da quella foto di gioventù morta per lavoro. Il mio foglio di appunti è bianco,

che sono la più alta forma di ingiustizia umana. Filippo, Marco e Roberto erano nostri fratelli, nostri cognati, nostri genitori, nostri figli: uno di loro aveva solo vent'anni. solo vent'anni. Dobbiamo fermare il Paese quando accade questo, ma non per commemorare, bensì per interrogare ogni giorno le nostre coscienze e fare quotidianamente qualcosa per evitare e scongiurare le morti sul lavoro. Abbiamo tre persone al giorno che escono di casa per lavorare e non vi fanno più rientro. Dobbiamo fermare il Paese per questo. Dobbiamo fare tanto, molto di più. Quanto ai abbiamo aumentato gli ispettori sul lavoro. Stiamo discutendo del superbonus: verifichiamo se la normativa sull'iscrizione delle aziende alla Camera di Commercio è corretta, facciamo tutto il possibile. Stamattina, un grande abbraccio e una immensa vicinanza alle famiglie di Marco, Roberto e Filippo per il loro dolore.

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 7 (rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2020) e 8 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2021). Il relatore, senatore Pesco, *relatore*. Signor Presidente, come ogni anno l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare gli atti relativi al bilancio interno dell'istituzione. Questa volta si tratta del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2020 e del progetto di bilancio relativo all'anno 2021 che il Consiglio di Presidenza ha deliberato nella riunione dello scorso 14 dicembre. Limitandomi a un esame essenziale di questi due documenti contabili e iniziando dal rendiconto relativo allo scorso esercizio finanziario, osservo innanzitutto come la spesa complessiva effettiva (al netto dei risparmi da versare allo Stato)

Va inoltre considerato che questo dato di riduzione della spesa, essendo espresso in termini nominali, non tiene conto della dinamica inflazionistica e dunque risulterebbe ancora più marcato, ove venisse espresso in termini reali. Peraltro, le entrate del Senato evidenziano che la dotazione finanziaria è rimasta invariata dal 2012 nella misura di circa 505 milioni di euro. Per conseguenza, rispetto alla dotazione richiesta nel 2011, pari a euro 526.960.500, si registra una riduzione annua di 21,6 milioni di euro. La costante riduzione della spesa negli ultimi anni si è dunque accompagnata a una sostanziale stabilità grazie a tutti contro il 45,41 di quella previdenziale, mantenendosi sostanzialmente costanti tali due elementi nel corso degli anni. Per quello che riguarda il bilancio di previsione 2021, oltre al dato già evidenziato della minor dotazione richiesta anche per l'anno in corso, si registra, per quanto riguarda le spese di natura previdenziale, un leggero aggiustamento per l'anno in corso rispetto all'anno precedente (in diminuzione per lo 0,09 Tuttavia, va rilevato che tale importo comprende anche le somme accantonate a seguito delle riduzioni introdotte sia per i vitalizi dei senatori sia per i trattamenti pensionistici dei dipendenti. In particolare, si evidenzia che i risparmi dovuti all'applicazione della riforma del calcolo dei vitalizi approvata nel corso dell'anno 2018 sono stati lasciati in un apposito fondo istituito prudenzialmente fino alla fine dell'*iter* processuale in corso presso gli organi di giustizia interna. Anche per quanto concerne l'applicazione del comma 261 della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a determinati importi annui lordi, si è proceduto all'istituzione del fondo del risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato, così come stabilito dalla stessa legge al comma 265. inoltre evidenziare la circostanza che nello scorso esercizio finanziario la spesa corrente obbligatoria ha rappresentato ben il 91,20 per cento di tutte le spese del Senato. Tale aggregato risulta in diminuzione da anni e comprende i risparmi e i costi per senatori ed ex senatori, personale di ruolo, in quiescenza o estraneo all'amministrazione, nonché tutti gli oneri collegati, quali quelli fiscali e previdenziali. Si registra altresì una leggera diminuzione nel triennio 2018-2020 anche per quanto riguarda la spesa corrente di funzionamento in senso stretto. Tale aggregato si compone di tutte le spese sostenute per l'erogazione di servizi e forniture di supporto al funzionamento del Senato, quali le prestazioni professionali per l'amministrazione, le spese per attività delle Commissioni, i costi per i servizi informatici, di comunicazione, assicurativi, ristorazione, trasporto, locazione, pulizie e altri. Risulta altresì in diminuzione la spesa in conto capitale tra il 2018 e il 2020, il 2020, che è passata da circa 2.465.013,75 euro a 2.277.204,10. La spesa in conto capitale, che costituisce l'aggregato meno rilevante in termini assoluti tra quelli precedentemente citati, comprende le spese per l'acquisto di beni mobili inventariati, le spese di manutenzione straordinaria, nonché quelle di acquisto e conservazione del patrimonio della biblioteca e dell'archivio storico. A fronte di una così marcata riduzione, le spese come quella registrata a partire dal 2012, la sfida è stata ed è tutt'ora quella di rendere compatibili i risultati finanziari conseguiti, che testimoniano la partecipazione del Senato allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica compiuto negli ultimi anni, con il mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dei servizi erogati, tanto più in un contesto che ha visto, almeno fino alla fine del 2020, una costante riduzione del personale di ruolo dell'Amministrazione.

Signor Presidente, ringrazio il presidente Pesco per la sua illustrazione. Cari colleghi, quest'anno ci apprestiamo ad approvare il rendiconto delle entrate e delle spese del 2020 e il bilancio interno del Senato per il 2021.

Grazie *in primis* ringraziare il dottor Marini, con cui abbiamo cercato di dare maggior sicurezza ai senatori, ma anche a tutto il nostro personale interno e a tutti i collaboratori,

di operare per il bene comune e per rendere sicuro il nostro Senato della Repubblica e credo che ci siamo riusciti.

dello Stato. Sul versante delle entrate, si è registrato un risultato complessivo nel 2020 pari a 542.905.117,10 euro. Grazie

Come si evince dai dati del rendiconto, l'azione di contenimento della spesa riguarda tutti gli ambiti della macchina amministrativa e credo che questo sia un altro aspetto fondamentale. Il rapporto tra spese di funzionamento e spese previdenziali

Mi fermo qui per quanto riguarda il Rendiconto e passo al bilancio di previsione 2021 che, come sapete, rispetto al bilancio provvisorio approvato a dicembre dal Presidente del Senato non presenta alcun tipo di variazione. Anzi, la validità tecnica e finanziaria e i numeri sono decisamente uguali a quelli attuali. Le riduzioni della spesa del 2021 per il funzionamento della macchina amministrativa un importo stimabile pari a 12 milioni di euro. Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto dal 2013 al 2021 di un importo pari a 322,5 milioni di euro. Ciò è stato reso possibile da una minore dotazione

difficoltà. Molto personale è andato in quiescenza e non abbiamo più avuto concorsi. Finalmente sono ripresi i concorsi con l'anno 2021-2022, sia per quanto riguarda i coadiutori parlamentari, sia per gli assistenti parlamentari.

delle aule di tutte le Commissioni con i sistemi di videoconferenza. È stata finalmente informatizzata la procedura di scrutinio del voto di fiducia, come avete visto negli ultimi In primavera sarà ammodernato l'impianto audio-video della 4a Commissione, che è l'ultima mancante in questo percorso.

la possibilità di accesso anche alle persone con disabilità. Particolare cura abbiamo dedicato al miglioramento dei ricambi

con tecnologie di virtualizzazione e tecnologie *cloud*, che ci permettono di lavorare a distanza. Il rinnovo di queste infrastrutture, che tengono conto anche degli aspetti *green* rispetto ai consumi, ci ha dato la possibilità di un risparmio di 15 milioni di euro

"Tabulas", che consente ai senatori di accedere ai documenti parlamentari, l'*app* "Senato Media" e una serie di altri interventi che stiamo facendo,

Infine, abbiamo lavorato sull'implementazione della *web* TV del Senato, con sette canali in contemporanea. Un altro aspetto su cui la collega Bottici si sta impegnando in maniera importante

al presidente Calderoli, che è oggi qui con noi, e a tutti i colleghi. Poi vorrei fare a tutti voi veramente un augurio di buon Natale e di buon 2022, a ognuno di voi: alle vostre famiglie e ai vostri cari a tutto il personale del Senato, che in questo ultimo anno è stato a sua volta attento, assieme a noi, per rendere la vita migliore possibile, a partire chiaramente dal segretario generale, la dottoressa Elisabetta Serafin, che ringrazio di cuore; ai vice segretari generali,

infine, non di certo ultimi per importanza, ai nostri assistenti parlamentari, che garantiscono in Aula la sicurezza e all'interno del Senato tutte le procedure che tutti noi conosciamo. *(Applausi)*. Quindi grazie a tutti voi

le spese ordinarie della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato sono state confermate: questo ovviamente è fonte di soddisfazione. La più peculiare delle competenze della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio storico, da me presieduta, però, è redigere il piano editoriale del Senato. Lo abbiamo presentato nel giugno 2019, ma l'organo investito della sua approvazione, il Consiglio di Presidenza, non lo ha ancora esaminato. Entriamo nell'ultimo anno di legislatura e la stampa di discorsi parlamentari come quelli di Banfi, di Cossiga, di Alma Capiello ancora non è potuta avvenire, in ragione di questo adempimento mancato. I Questori sono stati espliciti, sin dalla scorsa legislatura (XXI Collegio, 19 giugno 2014), sulla necessità della gara per l'individuazione dell'editore con il quale instaurare il rapporto di coedizione avente ad oggetto la pubblicazione dei volumi delle collane dell'Archivio storico. Ne deriva che, senza la possibilità di proroga dei vecchi editori e con un bando ancora da approvare, l'attività editoriale dell'Archivio storico procede a stralcio, come per le ristampe che meritoriamente la Presidente ha richiesto per Angelina Merlin o che noi abbiamo disposto per Emilio Lussu o Araldo di Crollalanza, utilizzando collane esterne. Altra modalità di intervento suppletivo è la coedizione con soggetti esterni, che, partecipi del progetto culturale di valorizzazione di documenti del nostro Archivio, si dichiarano disposti a scegliere e pagare l'editore. Abbiamo proposto la convenzione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, ma la trattazione in Collegio dei Questori è stata rinviata. Spero che venga ripresa quanto prima, in modo tale da consentire questa importante edizione. Lo proporremo di nuovo per il volume sui senatori del regno ebrei,

Altra conseguenza del blocco del piano editoriale è stata che ovviamente una delle risorse umane dedicate, con grande apprezzamento, all'attività di redazione dei discorsi parlamentari è stata distolta e inviata altrove, aggiungendosi ai molti segretari che, assunti come archivisti storici, svolgono mansioni in altri settori dell'amministrazione. Questo mentre la progressiva apertura alle desecretazioni, avvenuta nel luglio del 2020 con il decreto del presidente del Senato, comporta la gestione, nella nuova banca dati dell'Archivio, di oltre un milione di immagini scansionate soltanto per la Commissione stragi. Di qui la mia richiesta che nella prossima batteria di concorsi si contempli anche la professionalità archivistica o comunque una modalità per ricostruire il numero iniziale di unità dell'epoca della presidenza Pera. Non tutto comunque dipende da noi; anche se riuscissimo ad esitare in tempi celeri la richiesta di desecretazione di 130.000 pagine provenuta dall'onorevole Casson, la modalità ordinaria di attivazione degli interpelli appare vistosamente inadeguata. Ecco perché attendiamo dalla Presidenza del Consiglio risposta alla proposta di una nuova e più agevole modalità di esame delle richieste di declassifica. Nel frattempo, abbiamo dato istruzioni di dare attuazione in Senato all'ordine del giorno approvato in 7a Commissione il 23 novembre scorso sul segreto archivistico. Ricordo poi che le ristrettezze di bilancio hanno indotto a remunerare solo con titolo onorifico di consulenti coloro che, dedicando tempo ed energie, aiutano chi versa fondi privati ad inventariarli per poi renderli consultabili secondo il sistema di gestione archivistico presente in Senato. Questa modalità, totalmente gratuita, ritarda il conferimento dei fondi privati all'utenza; andrebbe ripristinata pertanto da parte del Collegio dei questori la maggiore disponibilità che a questo scopo era dedicata nelle scorse legislature alla stipula di contratti di acquisizione a titolo oneroso. Per concludere, voglio spendere una parola sulla lapide apposta nel cortile d'onore; se la monarchia ha fatto l'Italia, la Repubblica ha completato il *pactum societatis* con la promessa di maggiore giustizia sociale. Ho chiesto ripetutamente e chiedo in questa sede un completamento iconografico di quel fronte del cortile con richiami della Repubblica e della Costituzione. Mi aspetto che i Questori si dimostrino sensibili a questa proposta e che vogliano imprimere nell'ultimo anno del loro mandato una svolta culturale alla loro azione. Per mio conto, la Commissione procederà, con i mezzi di cui dispone, a valorizzare i suoi fondi archivistici e quelli che in sinergia con altre istituzioni culturali sta contribuendo a rendere noti. È il caso dei processi matteottiani, il cui restauro da parte dell'Archivio di Stato di Roma sarà oggetto di una mostra che svolgeremo in Senato nella prima metà dell'anno prossimo.

Signor Presidente, l'ordine del giorno G3, che ho voluto sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, ha l'obiettivo di disciplinare il rapporto di lavoro tra i parlamentari e i rispettivi collaboratori per porre fine all'annosa questione dell'inquadramento contrattuale di questi ultimi. Nonostante le Camere mettano a disposizione di ciascun parlamentare somme destinate al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, all'interno del Parlamento si rileva che parte dei collaboratori non ha un contratto regolare e non sempre la gestione di tali rapporti di lavoro appare limpida. Ciò non è concepibile, sia per la dignità del lavoratore sia per la mancanza di trasparenza, richiesta invece al mondo politico e alle Istituzioni da parte dell'opinione pubblica. Non è previsto uno specifico inquadramento contrattuale e di fatto i collaboratori parlamentari vengono equiparati ai dipendenti di studi professionali. È necessario tutelare la figura professionale del collaboratore parlamentare, ancor di più dopo il taglio dei parlamentari, che produrrà un aumento del carico di lavoro per i singoli, attraverso una regolamentazione chiara e trasparente che determini il contenuto essenziale dei contratti stipulati sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello normativo. Rivolgo un invito ai senatori Questori perché avanzino in Consiglio di Presidenza del Senato una proposta per giungere al pieno riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare, prendendo come modello le soluzioni adottate da molti Paesi europei e dal Parlamento europeo, nel rispetto dei seguenti principi: la gestione amministrativa e finanziaria delle posizioni lavorative dei collaboratori parlamentari sia ricondotta all'amministrazione del Senato, ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata come termine massimo alla durata della legislatura e del mandato parlamentare; l'istituzione di una voce nel bilancio del Senato della Repubblica vincolata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari con contratto; l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive, mutuando quanto in uso per i collaboratori dei senatori facenti parte del Consiglio di Presidenza o dei Presidenti di Commissione, nonché la disciplina degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. autorevoli quotidiani nazionali chiamano in causa il Parlamento, i parlamentari e questa Istituzione, che discute un passaggio così importante. A proposito dei collaboratori parlamentari, ritengo che sia giunta l'ora di fare chiarezza su questo punto, facendo in modo che nelle istituzioni parlamentari non alligni nessuna forma di potenziale illegalità. dunque i senatori Questori, nei quali ripongo massima fiducia, a fare in modo che un'azione sia svolta per risolvere questo annoso problema. Mi auguro che possa esserci un percorso condiviso anche con la Camera dei deputati, che arrivi a dare finalmente piena dignità e riconoscimento a coloro che quotidianamente ci accompagnano nella nostra attività e nell'azione parlamentare.

assieme per dare un aspetto normativo che preveda che il rapporto di lavoro continui a intercorrere direttamente fra senatore e collaboratori e sia caratterizzato da una natura fiduciaria - chiaramente, perché così dev'essere

Al riguardo va subito precisato che la proposta in questione è già da tempo oggetto di attenta analisi da parte del Collegio, che è sensibile a questa problematica ed è convinto che una soluzione debba essere trovata dalla prossima legislatura, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio, poiché non si può sforare. Come dicevo prima, la questione è oggetto di esame anche presso l'altro ramo del Parlamento, dove pure sono stati presentati analoghi ordini del giorno. L'intenzione del Collegio è di ricercare una soluzione più idonea, di concerto con i colleghi della Camera dei deputati e del suo Ufficio di Presidenza, in maniera tale da rendere uniforme eventualmente l'intervento in questo

Signor Presidente, colleghi e colleghe, interverrò molto brevemente e lo farò per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI ai due provvedimenti: il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2021. Desidero in primo luogo ringraziare sia il presidente del Senato Alberti Casellati sia il collegio dei senatori Questori per l'ottimo lavoro svolto con dedizione e senso delle istituzioni. Tengo altresì a dare conto anche del processo e della strada intrapresa già da qualche anno per la razionalizzazione delle spese del Senato, ma soprattutto della qualità delle stesse, nel rispetto del principio certamente dell'economicità, ma anche dell'efficienza. La nostra è infatti un'istituzione che ha bisogno di funzionare al meglio per le competenze che ci vengono assegnate. Questo aspetto viene in rilievo soprattutto sotto il profilo della razionalizzazione dell'attività amministrativa, al fine di raggiungere gli obiettivi che sono stati individuati in sede programmatica. Voglio sottolineare questo risultato a maggior ragione con riferimento al rapporto rispetto alla qualità della spesa. Vorrei soffermarmi in questa sede su due aspetti in particolare: un primo aspetto riguarda la significativa riduzione, come già avvenuto nel periodo precedente 2012-2019, della dotazione del Senato. La riduzione dall'inizio della scorsa legislatura è di oltre 190 milioni di euro. Questo *modus operandi* assume, a mio avviso, un significato importante: vuol dire che il contenimento della spesa non avviene in maniera sporadica, solo per quest'anno, ma sta assumendo carattere strutturale e sistematico. Questo aspetto non è di poco conto, posto che investe nel complesso l'intera Istituzione e riverbera i propri effetti anche al suo esterno. Strettamente correlata a questo specifico profilo, come sottolineato dal collega De Poli nella sua relazione, è la progressiva riduzione del peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica, frutto di scelte meritevoli, che sono state sviluppate in maniera costante nel corso di questi anni. Si tratta di un peso sulla finanza pubblica che si è ridotto in maniera considerevole (per più di 300 milioni di euro): più di 300 milioni di euro): questa riduzione, come già sottolineato, è, per l'appunto, il frutto di una serie di risparmi che sono stati effettuati nel periodo in questione. Il contenimento della spesa ha poi riguardato anche le indennità parlamentari e le competenze accessorie, con una diminuzione di 77 milioni di euro rispetto alla dinamica tendenziale. La percentuale della spesa per le indennità dei senatori rispetto al bilancio del Senato si è pressoché dimezzata, dal 2001 al 2021, passando dal 19 al 10 per cento. Infine, due note in merito ai fondi di riserva, l'uno obbligatorio, quello della legge n. 145 del 2018 per la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a determinati importi, che quindi va a costituire uno specifico fondo di risparmio, e l'altro riguardante le spese di natura previdenziale, in applicazione della riforma del 2018 per la riduzione dei vitalizi, istituito in maniera prudenziale e precauzionale in attesa che termini l'*iter* processuale interno agli organi di giustizia; mi sembra anche questa una scelta intelligente nella gestione finanziaria. Volendo brevemente entrare nel merito delle singole voci, mi soffermo unicamente su un aspetto. Si evidenzia come i principali scostamenti rispetto alle previsioni dell'anno 2020 siano il frutto di un aumento dello stanziamento resosi necessario per l'istituzione di nuove Commissioni d'inchiesta, per le quali, come sappiamo, le norme istitutive hanno previsto il relativo stanziamento di spesa a carico del Senato della Repubblica. Mi preme sottolineare

Consentitemi un'ultima osservazione. Lo sblocco del *turnover*, che avevamo tanto auspicato lo scorso anno, si è effettivamente verificato, pur nelle difficoltà che hanno caratterizzato le procedure concorsuali in questi mesi di pandemia. Mi permetto dunque di auspicare un'accelerazione di nuove assunzioni, affinché il personale dei nostri uffici venga supportato al più presto in modo adeguato e sufficiente a garantire una lineare attività per l'esercizio delle funzioni che che ci sono assegnate, quindi per dare il massimo dell'autorevolezza ai compiti che il Senato è chiamato a svolgere. Concludo il mio intervento con i ringraziamenti al presidente Casellati, al collegio dei senatori Questori. Ci tengo a ringraziare la dottoressa Serafin, che svolge il suo lavoro di Segretario generale con passione e dedizione, senza risparmiarsi mai, come anche i Vice Segretari generali del Senato. Desidero altresì ringraziare il dottor Sassoli per il suo prezioso e sempre attento contributo ai lavori dell'Assemblea. Un doveroso ringraziamento va anche ai direttori dei Servizi, ai funzionari di Commissione

pandemia. Un ringraziamento va anche ai Vice Presidenti che ci assistono sempre con pazienza. Infine, un grazie affettuoso a tutti i dipendenti e alle dipendenti del Senato per l'alto livello di professionalità

cercato di continuare a dare il nostro apporto al Paese, facendo quello che dovevamo fare. Credo che ci siamo riusciti in modo

a individuare le procedure che ci hanno consentito di frequentare in sicurezza il Senato. Spesso, quando parliamo della pandemia, ripetiamo la frase: «Niente sarà come prima».

ma ci ha portato a vivere un periodo di impegno istituzionale molto diverso e straordinario, tutto il Paese - è stato sottoposto ad un'attività di decretazione d'urgenza da parte del Governo che ha sostanzialmente modificato i tempi di lavoro della nostra istituzione e quelli dei senatori e dei Gruppi.

capire quali sono le condizioni che ci consentono di fare un lavoro istituzionale, parlamentare e politico di qualità in questa Istituzione. Da una parte c'è il tema della modernizzazione, della rifunzionalizzazione e della digitalizzazione, cioè di tutti quei presidi nuovi e dei dispositivi che dobbiamo mettere in campo per affrontare

direi quasi dogmatica. Oggi dobbiamo misurare i costi in funzione della qualità del lavoro. Ritengo che Ritengo che le risorse che dovranno essere destinate ai Gruppi nella prossima legislatura non potranno essere inferiori; so che è già stato aperto un tavolo

di riduzione dei costi e del numero dei parlamentari non può determinare una perdita di qualità

uscire dal binario del criterio della riduzione dei costi e passare su quello della qualità del lavoro che dev'essere svolto dal Senato, in condizioni anche difficili. Quest'anno abbiamo vissuto ritmati dall'uscita dei decreti-legge, avevamo tempi inferiori e spesso non abbiamo potuto sviluppare un'attività parlamentare normale, legata al bicameralismo (che vi ricordo esisterà anche nella prossima legislatura).

ci dobbiamo dare le risorse e l'organizzazione per lavorare qualitativamente in modo migliore, anche rispettando il il dettato costituzionale nella dinamica del rapporto che ci deve essere tra le due Camere. Non so quanto durerà

per far fronte e arginare la pandemia, continui e ci dia dei risultati definitivi e decisivi in tempi brevi. però, stiamo vivendo una situazione che non ci dà certezze per il futuro e, quindi, probabilmente dovremo continuare ad agire a fronte di provvedimenti che ci costringeranno a tenere ritmi serrati. Credo che questi siano tutti elementi che devono far riflettere noi, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori per immaginare un futuro cui, con numeri inferiori e con la riorganizzazione di cui si sta discutendo nella Commissione deputata, la situazione risulti affrontata in modo positivo ed efficace. Dobbiamo saper immaginare un modo di lavorare qualitativamente migliore di quello di quest'anno.

del Gruppo Partito Democratico sarà sempre positivo, costruttivo e a disposizione per sviluppare ragionamenti di intervengo sull'ordine i lavori. Abbiamo trascorso tutta la notte in Commissione bilancio. Siamo stati chiamati a votare il bilancio del Senato, ma adesso il presidente Pesco ci annuncia che in Commissione si torna a votare.

non è possibile sdoppiarsi. Cerchiamo di fare tutto; assecondiamo le tempistiche assolutamente senza precedenti di una maggioranza che fa votare per tutta la notte il bilancio dello Stato in Commissione,

nell'esprimere il nostro convinto voto favorevole come LeU-Ecosolidali, voglio ringraziare i senatori Questori e tutti coloro che nell'Amministrazione (i funzionari, gli impiegati e la Segreteria generale) si sono occupati del bilancio per il risultato raggiunto anche quest'anno. Non è mai facile tagliare i costi di un'azienda così complessa senza avere ripercussioni negative sulla vita e sulla qualità del lavoro dei dipendenti, siano essi personale amministrativo o senatori. I numeri parlano chiaro. E le giuste riflessioni del collega Collina ci impongono sempre di più, prendendo atto della necessità e dell'obbligo di convivere con questo convitato di pietra, con la pandemia,

Di questi, 194 milioni derivano dalla minore dotazione da parte dello Stato e 128 milioni da altri risparmi per il suo funzionamento. Negli ultimi quattordici anni il *trend* del rapporto tra la spesa effettiva del Senato e la spesa dello Stato è risultato sempre decrescente, passando dallo 0,083 per cento Il contenimento della spesa riguarda, in particolare, le indennità dei senatori e le altre competenze accessorie (meno 77 milioni di euro) e il loro rapporto con il bilancio del Senato, che risulta più che dimezzato negli ultimi vent'anni. C'è poi da considerare la riduzione della spesa per il personale, che ha portato a un risparmio di oltre il 22 numeri che risultano dall'opera di costante razionalizzazione dell'attività amministrativa in un'ottica di qualità, distinguendo sempre tra oneri di funzionamento, il cui contenimento della spesa è avvenuto in maniera trasversale, e oneri di natura strettamente previdenziale, che restano pressoché invariati. Ulteriori risparmi potranno derivare, per circa 12 milioni di euro per il 2021, dalle integrazioni delle amministrazioni di Camera e Senato, che hanno consentito la nascita del polo della documentazione parlamentare e del polo informatico parlamentare, oltre al rafforzamento del polo bibliotecario. Anche quest'anno l'azzeramento dei fondi di riserva pone una conferma sul tema della trasparenza, con tutte le uscite dettagliate voce per voce, pianificate, verificate, rendicontate. Gli scostamenti rispetto alle previsioni del 2020 hanno, in realtà, riguardato spese finalizzate a rendere il lavoro parlamentare ancora più efficiente e soprattutto più approfondito. Si tratta delle spese per le attività delle Commissioni di inchiesta, che sono aumentate di numero, e del necessario adeguamento delle strutture dei sistemi informatici. A ciò si aggiunge la locazione degli spazi necessari per lo svolgimento dei concorsi previsti per il 2021. C'è ancora da fare. Pensiamo soltanto alle opportunità di risparmio e di efficientamento in chiave ecologica, che derivano dall'uso delle tecnologie. Insomma, l'augurio è che anche i futuri risparmi possano coniugarsi con gli *standard* qualitativi che necessariamente deve mantenere

Ciriani, accertato che la sua richiesta non determina unanimità dall'altra parte, la Presidenza chiede alla 5a Commissione di sospendere le votazioni. Invito i colleghi che ancora devono intervenire in dichiarazione di voto di farlo nel minor tempo possibile, in modo da far proseguire i nostri lavori anche in 5a Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ritengo doveroso ringraziare il Collegio dei Questori, per il lavoro rigoroso e di qualità svolto fin dall'inizio della legislatura; il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti il Segretario Generale, dottoressa Serafin; il Vice Segretario Generale, dottor Toniato, e attraverso loro tutta l'Amministrazione, il Consiglio di Presidenza e tutto il personale, che quotidianamente operano con impegno per garantire il miglior funzionamento del sistema Senato. Un dato emerge dalla relazione del questore De Poli: dal 2013 ad oggi il Senato è riuscito a realizzare economie di spesa pari complessivamente a 322,5 milioni di euro, a riprova del grande equilibrio, della razionalità e del buon senso con cui è stata amministrata la Camera alta. *(Applausi)*. È bene ricordare che il lavoro svolto dal Collegio dei Questori ha due grandi obiettivi: garantire il miglior funzionamento della macchina legislativa, rendendo nel contempo la nostra istituzione, il Senato, una casa di vetro trasparente per i cittadini. Come abbiamo sentito, i numeri parlano chiaro: 194,4 milioni di minore dotazione da parte dello Stato dal 2013 ad oggi, a cui si aggiungono ulteriori risparmi pari a oltre 128 milioni, di cui una stima di 12 milioni di risparmi solo con riferimento al 2021. Sono la dimostrazione di come questa macchina amministrativa venga condotta con competenza e rigore, anche in un momento che è stato e continua a essere di grande difficoltà per tutto il Paese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A proposito di tutela sanitaria, il nostro pensiero va al dottor Federico Marini, che ringraziamo per la costante disponibilità e la preziosa competenza. Il Senato, infatti, anche nel cuore della pandemia, durante il *lockdown* dello scorso anno, non ha mai smesso di lavorare. I senatori Questori hanno saputo mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire - da un lato - la continuità dell'attività legislativa - dall'altro - la sicurezza sanitaria e la tutela della salute, a cui hanno contribuito parlamentari, personale e quanti fanno funzionare quotidianamente l'istituzione rispettando le regole. Il Senato ha dimostrato di sapersi adattare alla situazione emergenziale con tempestività, scelte strategiche e con investimenti anche tecnologici. La gestione del Senato si è dimostrata virtuosa, anche nella più difficile fase emergenziale in cui è stato più complicato riuscire a contemperare il doveroso risparmio con il buon funzionamento della macchina legislativa. C'è sempre il rischio, infatti, che, perseguendo l'obiettivo del taglio dei costi, si lasci indietro la qualità del lavoro, a maggior ragione nei momenti di crisi che hanno coinvolto e stanno purtroppo ancora coinvolgendo anche la gestione della nostra istituzione. I dati che sono stati richiamati dal senatore Questore anziano evidenziano, invece, che siamo in presenza di un'azione di attento monitoraggio dei flussi di spesa, decrescente nel tempo. Vorrei ricordare che la riduzione di spesa ha riguardato tutti gli ambiti della vita amministrativa e ricordo che, dall'inizio della scorsa legislatura, solo sul fronte delle indennità parlamentari e delle competenze accessorie, la stima delle economie di spesa si attesta su un importo pari a 77 milioni di euro, un cifra significativa. Come ho già sottolineato, però, ai cittadini interessano non soltanto i risparmi, ma anche l'efficienza delle nostre istituzioni. Per questo diventa importante migliorare e rendere più performanti i processi organizzativi interni. Penso - ad esempio - ai termini del pagamento delle fatture nei confronti dei fornitori, che avviene entro trenta giorni nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Penso al fatto che ridurre le economie di spesa vuol dire farlo con intelligenza e razionalità, non rinunciando quindi agli investimenti, con una prospettiva che sappia guardare al futuro. Per queste ragioni - come ha illustrato bene il senatore questore De Poli - noi riteniamo che sia stato importante e rilevante investire su fattori chiave come il digitale e l'innovazione tecnologica: il rinnovo delle infrastrutture informatiche ha portato a un risparmio pari a 15 milioni di euro, senza dimenticare gli aspetti fondamentali come le politiche *green* - lo abbiamo sentito - l'attenzione all'ambiente, il contrasto alle barriere architettoniche; quindi tutti gli interventi realizzati per

e per il mondo della cultura, che ha visto la nostra istituzione aprirsi ad eventi e incontri mensili promossi dal nostro presidente Alberti Casellati. Nel prossimo futuro ci aspettano dei cambiamenti radicali, a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari e, di conseguenza, del numero delle Commissioni e delle competenze del Regolamento. Si andrà verso una nuova disposizione per il Gruppo Misto, con una maggiore corrispondenza tra liste di eletti e Gruppi parlamentari. E di tutto ciò il bilancio interno del Senato dovrà tener conto, affinché al risparmio continuino a corrispondere l'efficienza e l'efficacia dell'azione legislativa, nonché di rappresentanza e di collegamento ancor più dinamico tra le due Camere. un percorso impegnativo in cui sono già coinvolti i nostri Questori in quest'ultima parte di legislatura. Li ringraziamo ancora per il lavoro svolto e per quanto continueranno a fare in questo passaggio molto delicato e complesso. Questore anziano De Poli, questore Bottici, questore Arrigoni, grazie per il lavoro e la disponibilità nel risolvere i piccoli e grandi problemi della vita di tutti noi nell'istituzione. Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC voterà convintamente a favore del rendiconto 2020 e del progetto di bilancio interno del Senato 2021.

brevissimo. Siamo consapevoli che anche per il 2021, come per lo scorso anno, l'attività del Senato è stata caratterizzata e influenzata dall'emergenza sanitaria Covid-19, che ha portato a modificare l'organizzazione dei lavori, ad accelerare sull'innovazione e sulla digitalizzazione e a spostare molte attenzioni ed energie dalle attività ordinarie verso quelle straordinarie e impreviste. Ricordo l'introduzione dell'obbligo del *green pass* per accedere alle sedi del Senato a partire dallo scorso 15 ottobre e del *super green pass* a partire dal 6 dicembre, per la partecipazione a iniziative istituzionali e culturali, convegni e conferenze stampa. Certamente apprezziamo i numeri positivi contenuti nei documenti del bilancio. Per il funzionamento del Senato, dal 2013 a quest'anno, si sono spesi meno 322,5 milioni. La spesa effettiva di questo ramo del Parlamento è in continua diminuzione sul totale della spesa statale, arrivando allo 0,045 per cento (dato che si evince dal rendiconto 2020). Vi è un progressivo contenimento della spesa per l'indennità parlamentare di noi senatori che, rispetto al bilancio dell'istituzione a cui abbiamo l'onore di appartenere, è passata dal 19 per cento del 2001 al 10 per cento del 2021, pressoché dimezzandosi. apprezzabile anche il fatto che il dover affrontare l'emergenza Covid non ha determinato alcun sforamento delle voci di spesa del bilancio, il che - soprattutto in questi due difficili anni trascorsi - è un segnale positivo e doveroso verso il sistema economico del nostro Paese in difficoltà, ma con gran voglia di ripartire nonostante le insidie del caro energia. Certo, giungere alla fine dell'anno, al termine dell'esercizio, a votare nell'Aula del Senato il bilancio di previsione 2021 è eccessivo, anche se so che il Collegio dei Questori lo aveva licenziato da tempo. Confido che il prossimo anno - per il quale tutti auspichiamo che i problemi e le conseguenze del Covid-19 per il nostro Paese si possano davvero attenuare - si possa procedere all'approvazione del bilancio preventivo nei primi mesi. Dobbiamo farlo per una questione di serietà dell'istituzione che rappresentiamo, visto che amministriamo soldi pubblici e soprattutto per il rispetto che dobbiamo ai cittadini. Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, non prima però di ringraziare il Collegio dei Questori e soprattutto il personale dell'amministrazione del Senato, a partire dal Segretario generale,

dall'inizio dell'emergenza Covid, ha messo in atto molte misure per contrastare il *virus*, garantendo - da un lato - la sicurezza sanitaria per prevenire e controllare il contagio di noi senatori

Signor Presidente, ciò che ci accingiamo a votare è un progetto di bilancio interno che - come emerso dalla relazione dei senatori Questori - si pone in linea con il processo di razionalizzazione della spesa di questa istituzione, ormai in corso da diversi anni e volto a renderla più efficiente e meno costosa; una razionalizzazione della spesa che, per il secondo anno consecutivo, ha dovuto tenere conto della situazione pandemica e delle conseguenti regole di condotta e svolgimento dei lavori, tanto per l'Assemblea quanto per le Commissioni. In quest'ottica, l'incremento di spesa per i cosiddetti servizi informatici, necessari per rendere più sicure le nostre infrastrutture e di conseguenza il nostro lavoro, rientra appieno nella *mission* di rendere questa istituzione più efficiente, oltre che più moderna. Aver garantito il giusto compromesso tra attività in presenza e in remoto ha permesso di non perdere il contatto, indispensabile e insostituibile, con il Paese reale, permettendoci di continuare ad audire associazioni, comitati e rappresentanze, assumendo così decisioni con maggior consapevolezza. Per quanto appena esposto, vorrei ringraziare tutto il personale del Senato, oltre che il Collegio dei senatori Questori, per l'incessante lavoro svolto per l'organizzazione delle nostre attività e il loro svolgimento in sicurezza. Un personale ringraziamento vorrei rivolgere al dottor Marini, che in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, ha mostrato grande disponibilità e sensibilità nei confronti di tutti, indistintamente. Guardando nell'immediato futuro, sono tante le sfide in ambito organizzativo e regolamentare che dobbiamo continuare ad affrontare. Con il termine di questa legislatura, ordinario o anticipato che sia, il nuovo Senato sarà composto da un numero inferiore di membri, ma resteranno invariate le richieste di sviluppo, crescita e risoluzione dei problemi che arriveranno dal Paese e che sono alla base del nostro lavoro quotidiano. Un numero inferiore di senatori, quindi, dovrà sopportare un carico di lavoro pari o maggiore a quello che oggi condividiamo tutti. In quest'ottica, il 2022 è l'ultimo anno utile in cui possiamo intervenire, tanto in ambito regolamentare, quanto di bilancio, per garantire ai futuri senatori uffici e assistenti parlamentari in grado di affrontare con successo la delicatissima sfida. Concludo, signor Presidente, dichiarando il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle e ringraziando ancora una volta l'intero personale del Senato per il lavoro che svolge ogni giorno.

Anche Fratelli d'Italia apprezza l'andamento di questi anni di riduzione della spesa del Senato. Ricordo che, se la dinamica della spesa generale dello Stato avesse seguito quella del Senato, adesso avremmo problemi di sovrabbondanza e di sapere dove allocare i soldi in più che abbiamo risparmiato, anziché grazie a tutti un ulteriore sforzo, senza che ciò incidesse negativamente sul saldo del bilancio. Ciò che più conta, nonostante l'emergenza, è che il Senato abbia potuto continuare a lavorare. Ricordiamo sempre che, nonostante qualcuno avesse scritto diversamente, il Senato è una delle istituzioni che ha continuato a lavorare anche nel periodo di più forti chiusure, quando la maggior parte delle altre attività era

Tutto questo è stato possibile grazie, naturalmente, al grandissimo lavoro del personale del Senato, per cui un ringraziamento va al tutto il personale, in particolare al Segretario generale, dottoressa Serafin, e ai vice segretari generali grazie a tutti fare il proprio lavoro, importantissimo e fondamentale, affidatogli dalla Costituzione, con sobrietà ma con efficienza. Questo è il nostro primo compito e su questo ci concentriamo. E, grazie al supporto che ci danno le strutture, possiamo portarlo Rivolgo per ultimo un ringraziamento al dottor Federico Marini, medico anziano del Senato, che, seppure particolarmente sotto pressione nel periodo di pandemia, è sempre stato una grande risorsa per questa istituzione.

per fortuna - la maratona in Commissione bilancio e che quindi ci apprestiamo ad iniziare la discussione

Questo ci consentirebbe di guadagnare tempo, di non avere quei lunghi tempi di attesa che di solito si verificano quando si aspetta il maxiemendamento (questo lo dico per esperienza personale), in modo tale da

Presidente Romeo, mi sembra molto ragionevole la sua prospettazione, fermo restando che

minuti fa. Grazie all'aiuto di tutti, a partire dagli Uffici, siamo riusciti a concludere il lavoro in un tempo sufficientemente breve per rispettare gli impegni grazie a tutti

dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, definiti a livello macroeconomico dalla Nota di aggiornamento al Documento La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche i finanziamenti, i rifinanziamenti e la riprogrammazione di entrate e di spese. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024, disposta con il disegno di legge di bilancio, si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei finanziamenti, dei rifinanziamenti e delle riprogrammazioni contenuti nella seconda sezione. La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 146 del 2021, il cosiddetto decreto-legge fiscale. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 nel 2023 e al 3,3 nel 2024; quindi un po' più alto nel 2022 e progressivamente scende fino al 3,3, riportandoci ai valori pre-crisi. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 203 miliardi di euro a 180,5 miliardi nel 2023 e a 116,8 miliardi nel 2024. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280 miliardi nel 2022, a 245,5 miliardi nel 2023

Le spese - e questo è un dato sostanziale della manovra di bilancio - aumentano di circa 47,8 miliardi di euro

Nel complesso, le misure recate nel disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: riduzione della pressione fiscale e contributiva, crescita degli investimenti per lavoro e famiglia, riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, sanità, scuola e molti altri. Io mi soffermo soprattutto sui primi due, ovvero sulla riduzione della pressione fiscale e sulla crescita degli investimenti. L'articolo 2 è molto interessante perché reca i famosi 8 miliardi di euro utili a ridurre il carico fiscale. state, poi, definite, grazie a proposte dal Governo approvate in Commissione, le innovazioni sulle aliquote fiscali per il prelievo, che hanno ridotto il peso fiscale per gran parte dei cittadini italiani; tratta della famosa riduzione delle aliquote, cui poi si è aggiunta una riduzione del carico contributivo per molti cittadini nelle fasce di reddito più basse. L'articolo 3 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*, istituite dalla legge di bilancio 2020. L'articolo 4 riduce l'IVA sui prodotti igienici femminili. L'articolo 5 modifica la *governance* sul fronte delle entrate in riscossione: è molto importante per riuscire a migliorare il rapporto tra L'articolo 6 è molto importante perché riporta l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità *online*.

tra cui molti di noi, sono rimasti perplessi perché il superbonus veniva un po' depotenziato, ma grazie all'intervento che siamo riusciti a fare in Commissione lo abbiamo riportato a livelli adeguati, soprattutto per ciò che riguarda la durata. È stato esteso, per tutto il 2023, anche alle case unifamiliari, è stato tolto il tetto dell'ISEE, è stato tolto il vincolo della prima casa per le case unifamiliari, è stato tolto il vincolo della CILA, che doveva essere presentata nell'anno scorso. Insomma, siamo riusciti ad apportare tantissime innovazioni, che consentiranno a molti cittadini che hanno una casa unifamiliare di fare i lavori. L'unico vincolo un po' stringente - dobbiamo ricordarlo - è quello di riuscire a fare almeno il 30 per cento dei lavori entro giugno 2022. Sappiamo che le aziende sono già piene di lavoro e che ci sono pochi ponteggi; però diciamo che, se una persona è in gamba e si affida a tecnici competenti, probabilmente riuscirà a iniziare i lavori e a efficientare la propria casa dal punto di vista energetico attraverso il superbonus 110 per cento. L'obiettivo finale di questa misura è riuscire effettivamente a inquinare meno, bruciando meno combustibile per riscaldare la propria casa; è un obiettivo compatibile con tutti gli obiettivi internazionali ed europei di riduzione delle emissioni gassose in atmosfera per contrastare il cambiamento climatico. Questa è una cosa molto importante. Passiamo all'articolo 10, che disciplina il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo; esso è molto importante per la transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica 4.0 e per altre attività innovative. L'articolo 11, molto importante anche questo, reca l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione di contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata Nuova Sabatini, importantissima per chi ha un'azienda, perché permette di innovarsi scaricando un po' degli oneri di finanziamento sul pubblico, nel senso che viene pagata una parte degli interessi per i finanziamenti, che è una cosa molto importante. molto importante. L'articolo 12, molto importante anche questo, prevede i seguenti interventi: la dotazione di un fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, mentre la dotazione del fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro. perché le nostre aziende hanno bisogno soprattutto di strutturarsi, per presentarsi meglio sui mercati esteri e per offrire i loro prodotti e i loro servizi in modo adeguato, soprattutto per quanto riguarda la concorrenza con le aziende estere. Mi fermerei qui. qui. Ho fatto un piccolo *excursus* sulle misure economiche e finanziarie a vantaggio delle famiglie, per quanto riguarda l'ecobonus, e delle imprese. C'è molto altro nel disegno di legge di bilancio. Siamo in tre, quindi ognuno di noi parlerà un po' di misure diverse. Siamo qui per ascoltare ciò

per decidere sul prosieguo dei lavori, fermo restando che, sulla proposta se concludere la discussione generale nella serata avanzata o se invece proseguire domani mattina, sono sempre in attesa che i Capigruppo si sentano e ci facciano pervenire una proposta condivisa. Sul prosieguo dei lavori la Presidenza fa sapere che è convocata una Conferenza dei Capigruppo domani.

forse più che in altri anni, la sessione di bilancio è stata frenetica, dati i tempi dei lavori che la Camera e il Senato si sono trovati ad affrontare. Quindi, la contemporaneità

i normali ritmi. Devo dire comunque che, insieme ai colleghi relatori, il presidente Pesco e l'esperto senatore Errani, abbiamo cercato di organizzare un lavoro ordinato che, proprio per la composizione della maggioranza di quest'Assemblea, ha visto un contatto continuo con tutti i Gruppi proprio per cercare di addivenire a risultati comuni su temi importanti.

elemento molto importante; il terremoto in qualunque legge di bilancio rimane sempre un nodo da sciogliere, un argomento sul quale lavorare parecchio, ma anche aspetti legati alla salute della persona, alla violenza, alle necessità che questa pandemia ha messo in evidenza: la sofferenza delle persone, degli adulti ma anche dei più piccoli e dei ragazzi, con tutte le varie sfaccettature che

però consentito di arrivare a interloquire con il Governo con molta determinazione. La cosa più importante era

devo dire che il *Premier* e il Governo tutto hanno dimostrato attenzione. Talvolta si dice che non è mai abbastanza, perché purtroppo i costi sono sempre altissimi, però è stata chiara la scelta di aiutare le famiglie, soprattutto quelle più deboli, a non soccombere travolte dal peso dei costi fissi di casa.

soprattutto ai commercianti e a tutti coloro che utilizzano spazi esterni, di essere aiutati

c'è chi dice che al Sud c'è una temperatura e al Nord è molto più difficile, però questa è stata una scelta che abbiamo fatto praticamente all'unanimità. Come dicevo, tanta attenzione è stata riservata alle persone e alle famiglie. Bello leggere dei giovani: ci sarebbe piaciuto avere molte più risorse per poter aiutare a nostra volta in modo significativo anche i giovani,

limitati, ma soprattutto limitati dalle scelte comuni che erano state fatte. In ogni caso, siamo andati avanti e abbiamo lavorato in questo modo. Secondo me è importante vedere come nasce un'idea di famiglia e come sia chiaro a tutti che si debba cercare di aiutare le persone ad essere famiglia, ad aiutarsi, a creare delle realtà di sicurezza e di crescita comune.

coinvolte e possano vivere in un contesto maggiormente inclusivo. Ad esempio, sono stati dati fondi ai Comuni per coprire i costi del trasporto

delle località turistiche da parte dei disabili. Questo ha una duplice valenza: è una platea particolare, ma è una platea che merita di vivere dei momenti felici in posti belli, magari anche facendo sport. Questo vuol dire cercare un modo migliore di vivere,

abbiamo già come base un Paese straordinariamente diverso e bello, ma dobbiamo imparare a farlo conoscere, farlo desiderare e renderlo

con l'Ape *social* a trentadue anni, a pensare a quei lavoratori che, facendo un lavoro molto usurante, hanno bisogno di

perché riuscire a coinvolgere queste persone, renderle più autonome possibili, vuol dire permetter loro di pensare ad un progetto di vita più sereno,

che ci sono in Italia. È incredibilmente straziante pensare che ci siano così tanti bambini sotto i sei anni che vivono nella povertà. Saremo più civili quando riusciremo quando riusciremo a migliorare la vita anche di queste fasce così deboli e troppo spesso misere non soltanto per mancanza di beni e di denari ma anche di

a cominciare dal fatto che il disegno di legge di bilancio è arrivato con oltre un mese di ritardo, per la scelta del Governo di mettere emendamenti pesanti dentro la legge di bilancio la maggioranza si avvicina sempre di più alla scadenza presidenziale.

che si è sviluppato tra i relatori, il Governo e i diversi Gruppi, compresi i Gruppi della opposizione, che per la loro la loro disponibilità a costruire questo dialogo credo sia giusto ringraziare. Abbiamo cercato di migliorare una manovra già espansiva. Il presidente Pesco ha spiegato i dati più ampi di macroeconomia: il legge di bilancio si colloca in una fase delicata di crescita che - non dovremo mai dimenticare - è inaspettata anche per noi

cui non sempre riusciamo a cogliere la profondità. Non di rado siamo autoreferenziali e pensiamo che la bandierina su questa o quella questione possa rappresentare parte di una risposta al Paese. Io credo, che siamo di fronte alla necessità di fare un salto di qualità nella capacità - e in questo il PNRR è importantissimo non semplicemente di fare le opere, non semplicemente di investire le straordinarie risorse contenute ma di definire un profilo nuovo di questo Paese. Noi siamo di fronte a cambiamenti inediti, che mutano l'antropologia di questo Paese. Il Covid-19, per me, ha certamente cambiato l'antropologia di questo Paese e dobbiamo fare i conti con sfide inedite per ampiezza e profondità, come la transizione ecologica, la crisi climatica, la rivoluzione tecnologica che produce sempre nuove forme di analfabetismo, di separazione e di frantumazione della società.

e sensibilità possiamo sottolinearlo, anche grazie al lavoro che abbiamo svolto in Commissione, scegliendo alcuni temi. quella di continuare a pensare che il superbonus non sia semplicemente un intervento per

Per questo abbiamo fatto alcune scelte importanti, come, ad esempio, la scelta irrinunciabile del fotovoltaico, senza

quella di dire che la transizione ecologica non è una scelta reversibile e che, anzi, dobbiamo costruire molto di più perché essa non sia reversibile.

troppo poco. Parliamo troppo di incentivi e troppo poco del nuovo progetto industriale di questo Paese. Forse questo è un limite di questo disegno di legge di bilancio, che o si incrocia con le strategie del PNRR, che guardano e vanno in questa direzione, o su questo avrebbe

proposito voglio esprimere una opinione strettamente personale che non riguarda in nessun modo gli altri relatori, che ringrazio per il lavoro importantissimo che hanno svolto.

Banca d'Italia parla di 109 miliardi di evasione fiscale, ma è difficile trovare un evasore, non perché non lo si trovi, ma perché nessuno pensa di esserlo:

a spiegare perché non siamo sempre dalla stessa parte, perché c'è una parte e perché ce n'è un'altra, in relazione alla strategia, alla visione, a dove si vuole portare questo Paese e i suoi cittadini, né sopra, suoi cittadini, né sopra, né contro di loro, ma neanche alla ricerca di un consenso effimero, giocato sul solleticare tutte le forme di egoismo.

allora come interpretiamo in forme moderne la redistribuzione, dentro a una inedita dinamica di accumulazione delle ricchezze. Io credo Io credo che nemmeno in epoche lontane l'accumulazione di ricchezza fosse così significativa come oggi,

di polemiche, tuttavia questa sintesi siamo riusciti a farla e la mettiamo a disposizione dell'Assemblea, dei Gruppi

Non voglio rinunciare ad affrontare questo problema. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che via via, diventando patologico, propone un problema significativo di di funzione non solo dell'Assemblea, non solo dei Gruppi, non solo del Senato e della Camera, ma della politica e non perché c'è Draghi, un tecnico, come Presidente del Consiglio. perché non riusciamo a sviluppare come dovremmo. Comincia a essere un problema confrontarsi e rapportarsi sulla dialettica tra tempi, tempo e possibilità di incidere, anzi di dire la propria. Questo è un grande problema. Non si può, l'ultimo mese prima del Natale,

perché in questo modo la politica perde di senso. Forse in questo difficile e a tratti anche abbastanza faticoso lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, con il

Prima di arrivare in Aula la manovra conteneva degli interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività.

per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come detto dai colleghi (che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare), ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità. Quindi questi sono i motivi per cui oggi si parla di espansività della manovra. Come dicevo, il lavoro della Commissione, sia per il tempo ristretto, sia per le forti divisioni di questa maggioranza, come faceva notare anche il collega Errani, forse perché si è alla fine di un percorso, non è servito, per quanto ci riguarda, ad apportare significativi miglioramenti al testo. Questo perché, si è letto e si è detto spesso - e non ho dubbi a confermarlo -, questa manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del *deficit* per 23,3 miliardi di euro. a quanto dicevo a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi che prima ricordavo: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità.

alla sua sospensione dall'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro. Voglio altresì ricordare

130 milioni di euro nel settore del *cross financing*. Per una partita di giro legata all'IVA, con questo emendamento, approvato grazie alla nostra sensibilità, ci sarà un risparmio di 130 milioni di euro.

ossia che serviva più coraggio. È vero, serviva più coraggio per fare questa riforma fiscale. C'è stato un taglio di 8 miliardi di euro,

Pertanto, sulla riforma fiscale, diciamo che va sempre bene quando si riducono le tasse, però questa riduzione varrà, come diceva qualche quotidiano nazionale, qualche caffè

200-300 euro l'anno, considerando che abbiamo inglobato anche i 100 euro di Renzi. Prenderemo quindi qualche centinaio di euro l'anno e ne perderemo 1.200. Effetti moltiplicatori con questa riduzione delle tasse purtroppo non ce ne saranno.

Pensavamo che potesse essere in qualche modo non dico stravolto, ma almeno cambiato; purtroppo questo non è accaduto. Il reddito di cittadinanza, come sapete, secondo noi, avrebbe dovuto essere una misura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché sappiamo che solo un terzo dei percettori del reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo diciamo noi, ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15

rispetto al testo iniziale effettivamente c'è un miglioramento. I lavori parlamentari sono riusciti, in questo caso specifico, a migliorare quanto era inizialmente previsto per il superbonus, eliminando dei paletti che il Consiglio dei ministri aveva messo nello schema di bilancio, che limitavano a tutto il 2022 la proroga del *bonus* per i lavori sulle case unifamiliari effettuati da persone fisiche. Effettivamente oggi con gli emendamenti vengono eliminati tutta una serie di paletti che creavano notevoli incertezze a questa misura. Ma, nonostante questo, va segnalata una tendenza che frena gli investimenti. Mi riferisco all'abitudine di cambiare le carte in tavola. Il superbonus, dalla sua entrata in vigore a oggi, ha già subito numerosi correttivi, che hanno in parte scoraggiato famiglie e imprese nello sfruttarlo per l'incertezza della sua validità, legata anche alle scadenze previste da una serie di misure. Rispetto ad altri temi contenuti nella legge riteniamo di essere in presenza di una manovra che non dà risposte né alle imprese, limitandosi a prorogare interventi già adottati negli anni passati, e neppure ai contribuenti, che continuano a essere perseguitati dall'Agenzia delle entrate. Voglio ricordare, una per tutte, le cartelle esattoriali, cioè le rate della rottamazione-*ter* del saldo e stralcio, che il 14 dicembre sono scadute; nessuno ha avuto il coraggio di intervenire almeno almeno per rinviare, in un momento delicato, questa misura così particolare. Proprio per questo dal Governo dei migliori c'era da aspettarsi una legge di bilancio ben diversa; non dovevamo certamente scomodare il presidente Draghi. Per quanto ci riguarda, questa è una manovra senza una visione politica, essendoci una maggioranza così eterogenea, che rinvia le scelte fondamentali e che dimentica totalmente la crescita. Un *iter* accelerato e allo stesso tempo frenato dai continui rinvii e dalle continue tensioni tra le forze di maggioranza ha evidentemente impedito di incidere e di migliorare questa manovra. Con questa breve relazione - chiaramente mi riserverò in dichiarazione di voto di fare un intervento prettamente politico - ho voluto motivare la valutazione contraria al testo approvato

Presidente, devo preliminarmente sottolineare alcuni aspetti che hanno caratterizzato la discussione su questa manovra. Nell'andare a sottolineare alcuni aspetti di metodo, voglio anche riallacciarmi a quanto detto poc'anzi dalla senatrice Rauti, che molto elegantemente ha rinviato a un altro momento qualsiasi tipo di ragionamento sul modo attraverso il quale si è arrivati oggi a discutere questa manovra di bilancio. Mi ha fatto piacere - lo ha sottolineato poc'anzi anche il collega Balboni il riconoscimento che ci è pervenuto, da parte del senatore Errani, sul ruolo responsabile che Fratelli d'Italia ha saputo svolgere all'interno di questo contesto. il fatto che ci sia stata riconosciuta questa dignità di opposizione responsabile non ci esime dall'esercitare la responsabilità anche nei confronti dei nostri elettori. Questo significa denunciare con forza il metodo adottato: mi riferisco ai continui rinvii che hanno caratterizzato la discussione di bilancio. La scorsa settimana la Commissione è stata convocata tre volte e tre volte quotidianamente è stata sconvocata. Siamo arrivati alla prima e unica riunione della Commissione bilancio, quella che si è svolta questa notte, che ha concluso i lavori e ci ha permesso finalmente di arrivare in Aula. Questo significa l'ennesima mortificazione nei confronti del Parlamento l'ennesima mortificazione nei confronti dell'unica opposizione presente in Parlamento, l'ennesima mortificazione nei confronti delle aspettative che tanti italiani avevano riposto negli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato in Commissione bilancio. Il fatto che ci sia riconosciuta questa dignità di opposizione responsabile non solo ci fa piacere, ma la rivendichiamo anche nel modo attraverso il quale il Gruppo si era organizzato, un modo che almeno personalmente ho condiviso e che credo, anzi ne sono sicuro, abbiano apprezzato tutti i colleghi parlamentari, perché siamo stati coinvolti tutti, a prescindere dai componenti della Commissione bilancio appartenenti al Gruppo Fratelli d'Italia. Permettetemi di esprimere dunque un sentito ringraziamento nei confronti del capogruppo Ciriani, del capogruppo in Commissione bilancio, senatore Calandrini, ma anche e soprattutto nei confronti dei colleghi parlamentari che hanno partecipato con attenzione, rigore e competenza a tutta la discussione preliminare che si è svolta all'interno del nostro Gruppo, che però non hanno avuto possibilità di esprimersi. Grazie anche al lavoro del gruppo legislativo e di tutta la segreteria del Gruppo parlamentare, abbiamo messo in campo una squadra vera che ha espresso o meglio avrebbe potuto esprimere in termini di competenza, un lavoro serio e approfondito. Questo non c'è stato consentito,

la *ratio* di ogni singola proposta emendativa presentata. Questo per quanto riguarda il metodo, ma ovviamente ci sono anche alcuni aspetti di merito che caratterizzano la nostra delusione. delusione. Mi riferisco in particolare a un comparto che non solo non è stato attenzionato nei giusti modi e termini, ma è stato addirittura vessato da

serie di misure negative che andranno a caratterizzare fortemente questo mondo. Ricordo che esso rappresenta all'incirca 20 milioni di italiani, con una percentuale importante del PIL sia per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo riferito al sociale, sia per quanto concerne lo sport, e che non è stato degnato della dovuta attenzione in questa manovra. In particolare c'è un provvedimento che grida vendetta, che è stato corretto in maniera parziale, andando a lasciare irrisolti i problemi che andrà a creare. Mi riferisco alla misura introdotta nel decreto fiscale, che andrà a modificare il campo di applicazione dell'IVA per quanto riguarda il mondo associazionistico. Un provvedimento pesantissimo, che è stato corretto solo parzialmente, utilizzando a mio avviso un modo di fare piratesco. La

Viene da dire che, tutto sommato, il problema temporaneamente è stato risolto. No, non solo è stato differito, ma addirittura ha aggravato la situazione di tutto il comparto.

riconosciuta dallo Stato italiano, che ha violentemente e pesantemente criticato questa manovra. Il provvedimento di rinvio non ha prodotto e non produrrà risultati efficaci. Il mondo delle associazioni infatti, che deve ancora cercare di capire se trasformare la propria natura giuridica da associazione semplice ad associazione di promozione sociale, andando a modificare il proprio statuto, con questa spada di Damocle rimasta sulla sua testa, non

in futuro si possa arrivare a una definizione, la più perentoria possibile, che risolva radicalmente la questione introdotta con l'approvazione del decreto fiscale. C'è poi un altro aspetto che

Da sempre diciamo che non ci potrà essere una crescita omogenea dello sport nel nostro Paese senza una sua crescita equilibrata all'interno delle nostre scuole. Ebbene, avevamo salutato con attenzione, curiosità e anche con rispetto

attenzione l'*iter* di questa parte della manovra. Purtroppo, questo aspetto legato alla possibilità di poter far finalmente crescere il mondo dello sport all'interno dell'istituzione scolastica è stato rivoluzionato, svuotato di significati e di investimenti, ed è stato ridotto a un mero provvedimento di facciata che andrà per l'ennesima volta a rinviare il problema. Ci sono anche altri aspetti che riguardano il mondo dello sport, un comparto che è stato lasciato ai problemi creati dalla pandemia e a quelli strutturali che riguardano tutto l'ordinamento sportivo, ma non è di questo che voglio parlare ora; ci sarà modo e possibilità di poterne parlare.

neanche di una discussione e che riguardavano la possibilità che le spese derivanti dalla crisi pandemica potessero essere affrontate con

da parte del Governo, ma anche del Parlamento, nei confronti di questa importante materia sociale. Già da ora segnalo e sottolineo il voto negativo di Fratelli d'Italia su tutta la manovra.

tra senatori, tra Gruppi e con il Governo, siamo qui a svolgere una discussione generale all'interno di un percorso di approvazione del lavoro importante fatto in Commissione. di legge di bilancio che già in origine era sicuramente molto espansivo: oltre 30 miliardi, di cui destinati alle spese sanitarie, 3 miliardi al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 3 miliardi agli ammortizzatori sociali, 2 miliardi e mezzo di interventi nel sociale, 2 miliardi per contenere i costi dell'energia, 1,5 miliardi per gli enti territoriali, 8 miliardi di riduzione di imposte, 2 miliardi di investimenti pubblici, 1,5 miliardi destinati direttamente alle imprese. Sono numeri assolutamente importanti di una manovra imponente, che aveva e ha il compito di iniettare in tutto il sistema economico di questo Paese una scossa importante e molto forte. In agricoltura, tema di cui mi occupo

citare l'esenzione Irpef, che vale quasi 250 milioni; la decontribuzione per gli *under* 40, che vale oltre 50 milioni in tre anni; l'intervento sull'IVA per la zootecnia da carne, che vale quasi 75 milioni; la gestione del rischio, che vale quasi 700 milioni in sei anni; l'intervento sulle assicurazioni, che ammonta a 250 milioni; l'intervento

2022-2023 e 40 a decorrere dal 2024; il tema delle filiere produttive, con 160 milioni stanziati per le filiere; i distretti del cibo (120 milioni); interventi sulla pesca; il fondo stesso sulla montagna: 100 milioni per molte aree rurali a più complicato contesto di sviluppo e a minore densità abitativa. Tutto questo a fianco degli straordinari interventi che stanno partendo per il PNRR, che inietterà quasi 7 miliardi di investimenti per logistica, meccanica, filiere, sistema irriguo e interventi di natura energetica.

dove, come è già stato detto dai relatori, sono state affrontate sfide molto importanti: interventi destinati alla scuola, alla cultura, all'ambiente, allo sport, alla ricerca, alle infrastrutture, al settore marittimo. Si sono affrontati temi delicati e molto complicati, come il tema cui si è fatto riferimento relativo all'IVA per il terzo settore, che nasceva da un rischio di infrazione comunitaria; la ridefinizione del *bonus* energetico; il tema molto delicato delle delocalizzazioni; questioni connesse alla libera professione. Ancora, il tema della riduzione fiscale e delle misure di natura previdenziale. Anche in campo agricolo si sono portati avanti interventi importanti a favore delle carni bianche, con un fondo che andrà a sostenere questo settore che sta attraversando oggettivamente una stagione di grande difficoltà generale legata, per certi versi, grazie a tutti

un provvedimento molto specifico sulla prevalenza, importante soprattutto in un'annata come quella che abbiamo alle spalle, con il gelo che ha colpito moltissime aziende. Si tratta del meccanismo di computo, secondo cui le aziende agricole devono avere prevalenza

straordinaria sia per le sfide che l'agricoltura, ma un po' tutta la società è chiamata ad affrontare in un momento di grande cambiamento, sia per le misure messe in campo. Come dicevo prima, tanti sono gli interventi sull'agricoltura; una stagione che vede all'orizzonte la nuova PAC e l'attuazione del PNRR con tutte le risorse e gli investimenti che andranno messi in campo. Una stagione straordinaria anche per le riforme che dovranno accompagnare il PNRR e che in agricoltura toccheranno tantissimi aspetti vitali: dalla digitalizzazione a tutta una serie di riforme organizzative di sistema; ma anche per il cambiamento di percezione che ruota intorno all'agricoltura. L'Unione europea, interpretando la sensibilità dei cittadini europei, ha recentemente approvato delle linee di indirizzo - dalla strategia Farm to Fork alla tutela della biodiversità che tendono a ripensare in una strategia di conversione l'agricoltura e il rapporto con il territorio in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale, di sostenibilità complessiva che guarda al futuro di queste produzioni. Sicuramente, come ho detto prima, l'agricoltura sarà chiamata a confrontarsi con una serie di sfide molto imponenti molto imponenti (la transizione digitale, energetica, ambientale), che richiederanno un cambiamento di paradigma organizzativo per certi versi, ma anche di ripensamento strategico delle propria finalità e modalità operative.

al tema della gestione del rischio, credo che questa legge di bilancio sarà ricordata nei prossimi decenni come quella che ha cambiato il sistema della tutela di fronte ai rischi catastrofali (gelo, siccità e alluvioni) per l'agricoltura, con un fondo mutualistico universale che andrà a sostenere

l'agricoltura sia chiamata nei prossimi anni e nei prossimi mesi a sfide molto importanti. Penso di poter dire che con questa legge di bilancio ci siamo corredati di una sorta di cassetta degli attrezzi che permetterà a tutte le istituzioni che lavorano a contatto con l'agricoltura di avere più strumenti cui attingere per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Ritengo che in questa legge di bilancio abbiamo fatto un passo importante. Sicuramente ci attendono impegni grandi nei prossimi mesi,

da un punto di vista parlamentare più anziana di me mi ha detto che neanche lei; un collega nei corridoi mi diceva che, con il tanto contestato Governo Berlusconi, si era alla presenza di signori. Credo che noi possiamo datare, dal 1994, una caduta libera per quanto riguarda questa istituzione parlamentare. Mi hanno raccontato che per modificare la Costituzione c'è un *iter* molto complicato

un *iter* che vuole custodire le regole parlamentari. Il Parlamento, oltre ad essere legislatore, anche se non lo è più da tempo, è anche controllore del Governo, ma neanche questo è più. Allora cos'è? Certo, con il taglio del numero dei parlamentari, con una legge elettorale che non verrà cambiata, perché non ci sarà il tempo,

è il partito a cambiare politica, il parlamentare è autorizzato, per il proprio mandato elettorale, a uscirne.

che non abbiamo. Infatti, 23,3 miliardi sui 37 sono a *deficit* e tra poco dovremo rendere conto di tutti questi movimenti a debito.

di presentare un decreto-legge che risolva la questione delle delocalizzazioni. Ebbene, la montagna ha partorito un topolino; anzi, ad ascoltare chi ha ben presente quali siano le conseguenze di questo emendamento del Governo, sembra che la pezza sia peggiore del buco, perché ponendo la questione soltanto in termini di pagamento, di prebende e di una maggiore multa,

tutto al *bon ton* istituzionale, andando a "sgridare" letteralmente quelle aziende che comunicano i licenziamenti con un sms. Eppure, una delle cose più importanti da fare è rivedere proprio la disciplina aziendale, secondo gli articolo 41 e 42 della Costituzione, perché non dobbiamo dimenticare l'articolo 41, al comma 1, prevede sicuramente che l'imprenditore abbia ragione e possa essere garantito nel suo *ius utendi*, ma al comma 2, laddove vieta un agire di impresa in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, nega lo *ius abutendi*. La conseguenza è che le imprese che intendono disimpegnarsi in via definitiva da un sito produttivo per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale, economico o finanziario possono venderlo ma non procedere alla sua chiusura. Eppure nessuna di queste procedure è prevista in questo emendamento. Nessuno dei subemendamenti all'emendamento del Governo, che prevedeva un

La visione del Governo, quindi, si può tradurre proprio in questa inadempienza grave nei confronti confronti delle delocalizzazioni. Un disegno di legge è stato scritto con costituzionalisti e tecnici del settore

senza ascoltare nessuna delle parti, è andato per la sua strada e, quindi, emetteremo multe che sarà facile pagare per chi vuole comunque prendere i soldi pubblici dell'Italia e poi andare a lavorare

abbiamo avuto prova di quanto il Titolo V sia stato deleterio e di quanto, invece che procedere sulla strada sbagliata, sarebbe necessario tornare a mettere mano al Titolo

sapevo che sarebbero arrivate le condizionalità, il cappio al collo per le città che sono state invece il bancomat dello Stato. La sottosegretaria

le critiche di metodo e di sistema, che mi auguro davvero che in questo ultimo anno di legislatura che ci attende possano essere corrette per consegnare alla prossima legislatura uno stile e una prassi parlamentare

una volta noi del Senato, una volta la Camera. Ciò di fatto pregiudica la ricchezza e la potenzialità del Parlamento.

nel disegno di legge e di ciò che diventerà operativo è quantomeno limitata dal tempo, se non dallo stato di vigilanza. La terza critica, che è la mia critica sistematica, mira a sottolineare come, con una maggioranza al 75 per cento dell'intero Parlamento, il ricorso alla fiducia sembra quasi un segno di sfiducia nei confronti del Parlamento stesso. Sono tre critiche di sistema, critiche procedurali che reputo importanti e che mi piacerebbe venissero ascoltate. Detto questo, quali sono gli aspetti che considero più interessanti e positivi di questa manovra di bilancio? Voglio soffermarmi, ovviamente, sul campo di nostra competenza, che è, al tempo stesso, un campo che riguarda la sanità ed uno che riguarda l'università. Per quanto riguarda il mondo della sanità, ho apprezzato molto l'aumento di due miliardi al fondo sanitario nazionale. Tanti o pochi che siano segnano, in modo in questo caso inequivocabile, l'inversione di tendenza, la considerazione che i costi per la salute non sono mai solo costi, ma sono sempre e soprattutto investimenti per la salute.

per sostenere gli ospedali che oggi si occupano dei bambini, che sono in questo momento la categoria più esposta. Bisognerebbe sentir parlare

Sostenere gli ospedali dei bambini diventa, quindi, in questo momento, la misura più coerente rispetto all'obiettivo che ci siamo dati. Mi rallegro anche perché è aumentato il fondo per i farmaci innovativi. Noi ci siamo rallegrati, poche settimane fa, per l'approvazione della legge sulle malattie rare. Abbiamo più volte sottolineato come una legge sulle malattie rare non possa essere efficace se non si sostiene la ricerca sui farmaci cosiddetti orfani e la sperimentazione che, mai come nel caso delle malattie rare, va verso farmaci innovativi, perché dobbiamo inventare farmaci che non esistono e non hanno un parametro di riferimento con altri. In questo contesto, mi rallegro anche di altre due misure. Una è l'aumento di 12.000 borse di specializzazione per gli studenti, per i giovani laureati in medicina. 12.000 borse in più significa in qualche modo recuperare quel *gap*, che era alle nostre spalle e che vedeva un imbuto che si stringeva e condannava in qualche modo, non alla disoccupazione, alla inoccupazione o alla occupazione meno qualificata tanti giovani medici, che comunque presentano un costo non irrilevante per la loro formazione. Lo stesso discorso vale per la stabilizzazione del personale assunto durante la pandemia,

sicuramente complessa e resa complicata dal contesto generale nel quale ci stiamo muovendo. Difficoltà anche a chiudere i conti, difficoltà a dare delle risposte complessive al Paese, che tengano conto di tutte le complicazioni che abbiamo davanti. Sicuramente il lavoro fatto dai relatori merita rispetto, attenzione e considerazione e in questo senso li ringrazio particolarmente. Non Non mi sento però di essere altrettanto generoso nei confronti del Governo, perché onestamente non è la quantità di risorse messe a disposizione che deve poi determinare l'applauso, ma la modalità con cui ci si rapporta per costruire una legge di bilancio importante. È evidente che stiamo facendo questo passaggio con tempi stretti e con difficoltà, come ha correttamente detto il senatore Errani, che ringrazio per l'attenzione particolare che ha messo su alcuni emendamenti relativi a Vigili del fuoco.

Penso a tutto quanto riguarda la riformulazione delle norme sulle tasse e la messa a disposizione, che abbiamo insistentemente voluto e sostenuto, delle risorse per poter

tuttavia anche tante misure minute, magari per qualcuno meno importanti, ma per noi davvero rilevanti, che abbiamo voluto sottolineare: in particolare, penso alle risorse messe a disposizione per le disabilità. Accanto a tutto questo, accanto a questi pesi massimi, ci sono poi questioni che non dobbiamo trascurare. Mi riferisco in particolare

di singoli senatori o di singole richieste del territorio, perché alla fine la narrazione esterna tenderà ad essere inevitabilmente quella di un Parlamento bloccato con settimane e giorni di lavoro (mentre il Governo è molto laborioso), per portare avanti delle piccole come vengono anche definite in termini tecnici. Questo non è corretto, perché il lavoro fatto in Commissione è impegnativo, difficile ed importante. Forse sarebbe meglio e più dignitoso ricondurre questo tipo di iniziative a un singolo provvedimento specifico: una volta la chiamavano in maniera dispregiativa «legge mancia», ma al suo interno si mettevano tante misure, magari anche l'intervento per sostenere una scuola o un'associazione, che è cosa differente rispetto ai macrocapitoli e ai macrotemi che devono invece entrare nella legge di bilancio. Oggi, il fatto di trovare mescolati questi due elementi sicuramente non rende un favore al Parlamento e non dà neanche l'idea della difficoltà del lavoro svolto e delle risposte

che abbiamo voluto insieme ad altri Gruppi e che il Governo ha consentito, con una riformulazione adeguata, di poter inserire nel disegno di legge di bilancio. Penso altresì alla riformulazione che ha raggruppato emendamenti fatti da più Gruppi che, come il nostro, richiedevano un rafforzamento degli organici dei Vigili del fuoco. Su questo bisognerà stare molto attenti perché è un meccanismo che pesca da un unico grande contenitore, all'interno del quale andranno a prendere le loro quote sia la Polizia di Stato che le altre polizie o i Vigili del Fuoco. Dipenderà dalla capacità che avrà il Ministero, e in questo senso saremo guardinghi, affinché non ci siano solo le briciole per i Vigili Fuoco, ma un significativo potenziamento del contingente di persone a disposizione.

Gli antichi dicevano «*pacta sunt servanda*»: si devono mantenere sempre gli impegni, al netto delle loro dimensioni. Se si manca nella parola, non c'è più fiducia. Chi rappresenta il Governo deve essere il primo a garantire il mantenimento della parola data nei confronti del Parlamento.

Questo avviene perché non si vogliono scontentare *lobby* o gruppi di potere. È negativo in questa manovra che gli uffici abbiano dovuto lavorare fino all'ultimo su emendamenti governativi che continuavano ad essere depositati, nonostante la contrarietà di tutti i Capigruppo; quindi gli uffici purtroppo non hanno avuto modo e tempo di completare tutte le istruttorie sugli emendamenti segnalati dai Gruppi. Come al solito, il Gruppo più sacrificato è stato il mio, il Gruppo di maggioranza relativa. Mi lasci anche dire, Presidente, che questo Gruppo però non è più disposto al sacrificio: dei nostri 140 emendamenti segnalati, quasi la metà purtroppo non vede la luce perché carente di relazione tecnica o di parere o di istruttoria. Eppure abbiamo lavorato per settimane, con grande impegno, per far sì che le poche risorse a disposizione del Parlamento fossero utilizzate in maniera efficace, provando a convergere su temi comuni. Le assicuro che in una maggioranza così variegata trovare la sintesi non è

le modifiche erano impossibili dato che il tempo era ormai scaduto. Quindi, Presidente, come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle mi lasci rappresentare oggi tutto il disagio che sta vivendo il mio Gruppo parlamentare. Mi lasci anche chiedere al Governo e ai dirigenti degli uffici ministeriali più attenzione per questo Gruppo parlamentare. Questa, però, è anche la manovra di alcuni *record* positivi e di questo parleranno i colleghi che mi seguiranno. Tra le cose positive certamente vi è la proroga dell'estensione del superbonus.

misure a sostegno della parità di genere e contro la violenza di genere, le misure a tutela degli animali, le misure in ambito sanitario, come l'istituzione del fondo per la genomica oncologica o dei disturbi alimentari, il fondo per la fibromialgia e, ancora, i tanti interventi a sostegno della ricerca. Qualcuno dei miei colleghi, però, evidenzierà anche le tante cose che purtroppo non siamo riusciti a fare. Non siamo riusciti ad erogare l'indennità di specificità agli infermieri. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma avevamo un parere contrario del Ministero della funzione della funzione pubblica. Non siamo riusciti ad estendere l'indennità prevista per gli operatori del Pronto soccorso anche agli operatori del 118: medici e infermieri sono stati i nostri eroi in questa pandemia, eppure ancora oggi non diamo risposte concrete a tutti.

Ce l'abbiamo messa tutta, però purtroppo queste battaglie non sono state condivise dagli altri Gruppi politici. Anche in questo disegno di legge di bilancio, nonostante le poche risorse, alcuni hanno preferito destinare i fondi ad interventi locali e - mi lasci dire - troppo territoriali, che dovrebbero essere finanziati in altro modo. Tra questi vi sono - cito solo degli esempi - il rifacimento del lungomare di Nicotera e i lavori di manutenzione della strada comunale per il mare o l'assunzione di due unità di personale per il Comune di Verduno. È chiaro, tutti i Comuni hanno bisogno di risorse. Noi avremmo voluto istituire un fondo proprio a supporto dei Comuni, per assumere più personale. Signor Presidente, il mio auspicio è quindi che questo Parlamento abbia una visione più ampia, che corrisponda al futuro di questo Paese. L'Italia è un grande Paese, gli italiani sono un grande popolo e la politica deve essere all'altezza del compito che le è stato affidato.

del principale Gruppo di maggioranza, che ha appena concluso il suo intervento. E devo dire che il Capogruppo del principale Gruppo di maggioranza sta rubando il mestiere all'opposizione, perché si è giustamente lamentato del fatto che questo Governo, il Governo Draghi, non ha innovato in alcun modo la prassi dei precedenti Governi, ma anzi l'ha aggravata, nella misura in cui i tempi a disposizione del Parlamento per esaminare un provvedimento importantissimo come la legge di bilancio non solo non sono stati dilatati, ma sono stati ulteriormente compressi, con la gara - aggiungo io - di tutti i Gruppi a portare a casa il loro piccolo risultato di campanile. Anche su questo faceva considerazioni assolutamente condivisibili la principale forza politica della maggioranza: ognuno porta a casa il suo piccolo risultato di cortile, di campanile, ma poi la visione complessiva rischia di essere persa o - peggio ancora - di essere imposta al Parlamento, che non ha più alcun margine per incidere sulle scelte importanti del prossimo anno, anno che sarà decisivo per la ripresa economica, ma anche per lenire le molte piaghe che la pandemia, da un lato, e l'inefficienza dei Governi che l'hanno dovuta affrontare, dall'altro, hanno purtroppo lasciato in tutto il Paese. Ebbene, cari colleghi, se questo è il giudizio della maggioranza, del principale Gruppo di maggioranza, che cosa dovremmo dire noi dell'opposizione? Dobbiamo dire che avete perfettamente ragione; che non si può continuare con fiducia su fiducia; che non si può continuare a mortificare l'Aula del Parlamento; che non si può continuare a trasformare il Senato, come del resto la Camera dei deputati, in una scatola vuota, priva di ogni valore. Ma vede, cara collega Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, tra noi e voi c'è una differenza: voi vi lamentate e rimanete esattamente al vostro posto a eseguire gli ordini che vi arrivano dall'alto; coerentemente di voi, rimaniamo all'opposizione e diamo il nostro contributo costruttivo quando veniamo ascoltati, le rare volte in cui veniamo ascoltati. di volte certamente ci siamo riusciti. Li citava prima il relatore di minoranza, il senatore Calandrini, che ringrazio,

per i proprietari di case che non riescono a rientrare in possesso del loro immobile: subiscono il furto del loro immobile, lo Stato non reagisce e non glielo riconsegna nei tempi dovuti. Abbiamo tenuto un fondo da 10 milioni per ristorarli e risarcirli. Voglio ricordare la battaglia importantissima per tutelare i professionisti che hanno un infortunio e si ammalano. Sono provvedimenti che Fratelli d'Italia ha fortemente voluto e che per fortuna si è riusciti a ottenere. Ma purtroppo, come Vice Presidente della Commissione giustizia del Senato, non posso tacere sul vergognoso emendamento riguardante la magistratura onoraria che il Governo ha appiccicato, quasi alla alla fine di questo pur modestissimo confronto, per far fronte alla procedura di infrazione annunciata dall'Europa nei nostri confronti, per il modo in cui l'Italia, in tutti questi anni, ha trattato e continua a trattare i magistrati onorari: trattati come veri e propri *rider* della giustizia, anzi peggio, perché adesso i *rider* fortunatamente verranno regolarizzati e stabilizzati. I giudici onorari - come sappiamo tutti benissimo risolvono quasi la metà di tutti gli affari della giustizia, la quale, senza di essi, semplicemente si fermerebbe. Senza i vice procuratori onorari non sarebbe possibile tenere udienza, e non dico davanti al giudice di pace, ma nemmeno davanti al tribunale; senza i circa 2.000 giudici onorari di tribunale sarebbe impossibile comporre una infinità di collegi. Sappiamo tutti molto bene senza i magistrati onorari, la giustizia domani mattina in Italia semplicemente si bloccherebbe. Si tratta di magistrati che, per anni, hanno lavorato senza tutele

qual è il riconoscimento, quale la gratitudine che il Ministro della giustizia e il Governo manifestano con l'emendamento citato nei confronti di questa categoria che ha tenuto in piedi la giustizia italiana?

al personale amministrativo, voi non offendete soltanto la magistratura onoraria, ma anche l'alta funzione giurisdizionale svolta in nome del popolo italiano. È una vergogna che in quest'Aula noi vogliamo denunciare in modo molto forte e chiaro. Come denunciamo l'illogicità, l'incongruenza e la contraddizione di pretendere di sottoporre a una prova selettiva con tanto di esame, seppur orale, magistrati

che il Governo doveva e poteva risparmiare a questi fedeli funzionari dello Stato. Caro Presidente, la cosa però veramente vergognosa è che con questo emendamento il Governo impone al magistrato, che dovesse accettare questa pur umiliante stabilizzazione, nel

diritti. Ai diritti che spettano a tutti i lavoratori, per il passato, deve rinunciare agli arretrati, ai diritti previdenziali e assistenziali. Deve rinunciare a tutto quanto. un ricatto imposto per legge che grida vergogna nei confronti di chi ha un minimo senso di giustizia. Ma quale Stato di diritto si comporta in questo modo nei confronti dei suoi fedeli servitori, come hanno dimostrato di essere i giudici onorari

disciplina molto delicata e importante della magistratura onoraria fosse stata affrontata e risolta nelle sedi opportune: la Commissione giustizia, prima, e l'Aula del Senato, poi, e ovviamente la Camera, dove si doveva affrontare non certamente sotto l'urgenza di una legge di bilancio ma - come voi stessi dite - con il tempo necessario con il tempo necessario per poter analizzare e discutere. Voi avete voluto chiudere ogni confronto, ancora una volta con un atto di forza, fregandovene dei diritti di una categoria di lavoratori così importante, collegata addirittura all'esito del PNRR. *(Applausi)*.

ringrazio anch'io i membri della Commissione bilancio, i relatori e il Presidente, che hanno lavorato alla difficile costruzione della legge di bilancio. Voglio partire anch'io - come hanno fatto la senatrice Castellone e il senatore Candiani - da un punto: è evidente che anche l'*iter* di questa legge di bilancio conferma che non può funzionare in questo modo. Non c'è solo un tema che riguarda il monocameralismo di fatto; non c'è solo un tema che riguarda l'emergenza costante con cui lavoriamo. È evidente

i grandi assetti, gli investimenti e un'idea di futuro del Paese, dobbiamo trovare il modo di evitare che questo procedimento vada insieme a un procedimento assolutamente legittimo, nell'ambito del quale i parlamentari cercano di portare avanti istanze o territoriali o di parte.

prima, per capire come si può impostare in maniera diversa la discussione e il lavoro sulla legge di bilancio. C'è una cosa a cui tengo, signor Presidente, e lo dico con forza a lei e alla Presidenza:

di alimentare un antiparlamentarismo di cui non c'è bisogno. Scaricare sul Parlamento e sull'istituzione tutte le responsabilità di quello che non funziona *(Applausi)* non credo sia accettabile, e credo che quest'Assemblea debba rispondere. debba rispondere. Nelle trasmissioni televisive di oggi, quasi ovunque i commentatori spiegavano che il Parlamento non funziona. Credo che le cose siano un po' più complicate e che alimentare l'antiparlamentarismo non sia utile.

si occupa davvero della salute dei cittadini stanziando grandi risorse sul tema della sanità in un momento così difficile di emergenza e di pandemia come quello mette in campo investimenti per aiutare la ripresa; aiuta i lavoratori e i più deboli della nostra società.

delle tasse sui salari dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; si è confermato il *bonus* dei 100 euro per i redditi fino a 15.000 euro; l'intervento sulle bollette aiuta soprattutto i più deboli; si interviene sulle due figure più penalizzate in questa società: i giovani e le donne. Credo che la norma sull'apprendistato, che esonera dai contributi, quindi ci porta a superare l'orribile pratica degli *stage* gratuiti, sia una misura importante; così come credo sia importante la norma

E lo abbiamo fatto con una maggioranza ampia, una maggioranza tra diversi, e rivendico

abbiamo cominciato a farlo con la pandemia perché prima non era così. Oggi i lavoratori autonomi e i lavoratori delle aziende sotto i 15 dipendenti potranno contare sugli ammortizzatori sociali, sulla cassa integrazione, sul sostegno nei momenti più difficili.

che, sulle questioni sociali e del lavoro, fa fare passi avanti rispetto alla riduzione delle diseguaglianze. poi la scelta del superbonus, la reiterazione, il sostegno, l'aumento delle risorse: è una straordinaria occasione per il Paese, per le aziende,

di incentivare tutte le aziende a innovare, perché pensare all'efficientamento energetico, alle tecnologie che servono per l'energia alternativa, per

con la forza di una capacità tecnologica e di innovazione mai avuta in passato. Ovviamente il superbonus vuol dire anche tutela dell'ambiente e della sicurezza del nostro costruito e significa, complessivamente, qualità sociale della città. Signor Presidente,

della magistratura onoraria, per dare ad essa risposte e certezze e superare la procedura di infrazione. Penso che il Governo, in piena autonomia, si sia assunto la responsabilità di scegliere come usare quelle risorse e ne prendiamo atto. Avremmo preferito anche noi che quell'emendamento venisse discusso col Parlamento, che stava lavorando da tempo sulla riforma, ma il Governo ha scelto un'altra strada. Avremmo preferito una strada che coinvolgesse il Parlamento: vediamo se quella strada produrrà l'effetto di superare il rischio di infrazione europea e se raccoglie le istanze delle associazioni.

all'inizio di questo dibattito - come ricordava il collega senatore Barbaro - ci avete riconosciuto la dignità di opposizione responsabile, che suona un po' come l'onore delle armi. Tale dignità di opposizione responsabile è dettata dal fatto che il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato oltre 700 emendamenti ragionati, di buon senso e propositivi al disegno di legge di bilancio, quando ancora speravamo di poter apportare

Forse ci riconoscete la dignità di opposizione responsabile per le nostre presenze in Commissione, naturalmente quando le sedute si sono svolte, perché - come sappiamo - la Commissione è stata continuamente sconvocata e paralizzata dai veti incrociati

per come arriviamo oggi fin qui e perché non si riesce mai a migliorare ciò che è più importante per la Nazione. E ce l'abbiamo messa tutta, dal buon senso, alla buona volontà. Ce l'abbiamo messa tutta, ma sbattiamo contro un muro di gomma e la sensazione, che riguarda tutti e non soltanto l'opposizione, è quella di un progressivo svuotamento

quanto segue: il 28 ottobre il Consiglio dei ministri adotta il disegno di legge di bilancio, che si presumeva sarebbe stato trasmesso al Senato in data 2 novembre. Come tutti sanno, non fu così e in quella *road map* si ipotizzava una possibile approvazione in prima lettura qui al Senato tra il 13 e il 17 dicembre e una possibile approvazione definitiva alla Camera tra il 20 e il 23 dicembre. Letta oggi la *road map* fa un po' ridere, se non addirittura piangere, perché questa è la storia. Com'è andata lo sappiamo bene e lo sento dire, tra l'altro, anche da esponenti della maggioranza. Evidentemente non siamo noi dei visionari negativi, morbosi e malati; anzi, noi abbiamo cercato di contribuire, ma la realtà oggettiva è spaventosa ed è quella che oggi qui, tra pochi intimi, ci stiamo raccontando.

Ne abbiamo fatto oggetto di un emendamento e poi di un ordine del giorno che è stato approvato in Commissione: mi sto riferendo alla nota *tampon tax*, ovvero all'articolo 4. È evidente che prendiamo atto che il Governo ha inserito nella legge di bilancio una significativa variazione dell'aliquota IVA, dall'ordinaria al all'agevolata al 10 per cento, per i prodotti dell'igiene femminile non compostabili, in quanto gli altri già godono di una IVA agevolata. Questo è in linea, tra l'altro, con la direttiva della Comunità europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che prevede che gli Stati membri possano applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, per la cessione di beni e prestazioni di servizi di alcune

di un riconoscimento, un sostegno, un aiuto e un segnale alle donne, in quanto si tratta di un bene - ripeto - necessario e non voluttuario. È uno sforzo che potete fare. Faccio presente che abbiamo fatto lo stesso ragionamento di abbassamento dell'aliquota e di aliquota agevolata al 5 per cento per i prodotti legati alla prima infanzia, che sono tantissimi e costosissimi, e ciò aiuterebbe le famiglie. Quando sento parlare di

sulla base delle reali esigenze della Nazione. Per esempio, Fratelli d'Italia ha chiesto di concentrare il taglio sul cuneo fiscale, sul costo del lavoro per sostenere le imprese. Abbiamo fatto delle proposte concrete e invece niente. Probabilmente la legge di bilancio è soltanto l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte con idee diverse che vogliono stare insieme e che, però, insieme non riescono

a fare nulla. Il compromesso al ribasso produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo patria.

mezz'ora fa della collega Nugnes sul tema. Non basta effettivamente fare una professione di intenti. Spesso e a tratti sentiamo degli interventi da parte del presidente Draghi o dal ministro dell'istruzione Bianchi o da altri esponenti del Governo. Ma, se di fatto non si pongono in essere delle soluzioni, è chiaro che rimangono parole al vento. In questa manovra con gli emendamenti abbiamo provato a dare una prospettiva in questa direzione. È importante in questo momento evidenziare anche un passaggio compiuto da un nostro europarlamentare, l'onorevole Procaccini, il quale proprio qualche giorno fa ha depositato una risoluzione per chiedere

come diceva la collega Rauti - che richiederà degli interventi a breve, medio e lungo termine. in Commissione europea è di destinare delle quote dei fondi dell'Unione europea agli Stati membri per far fronte a queste necessità. Come abbiamo visto dagli ultimi dati Istat, l'Italia

tenendo conto del fatto che, a livello europeo, la media è di 2,1 come soglia di sostituzione, per permettere appunto un ricambio generazionale.

da proporre per uomo e donna, ma noi sappiamo benissimo che, tra il compenso mensile di uomo e donna, c'è uno scarto di circa a discapito del sesso femminile. Quindi, è chiaro, a fronte delle opportunità, quale quella attualmente in vigore, del congedo parentale fino a sei mesi dell'età del bambino con una decurtazione dello stipendio del 70 per cento, quale dei due sessi farà maggiormente ricorso. Comunque, non è solo questo il punto. Il punto è anche legato a una esigenza di tipo pedagogico, alla crescita armonica, anche serena, del bambino e, soprattutto, a dare l'opportunità alle famiglie e alle giovani coppie di scegliere la soluzione più consona alla propria situazione di vita. A questo si potrebbe anche accompagnare - come molti hanno anche rilevato e come Fratelli d'Italia dice spesso - l'abbassamento del cuneo fiscale, ma anche un intervento per le piccole e medie imprese, e quindi per gli imprenditori, nel momento in cui

Perché non pensare - ad esempio - a una priorità per i giovani neolaureati o neodiplomati, che vediamo puntualmente migrare? Quando parliamo di inverno demografico, nell'immaginario collettivo ci si sofferma semplicemente sulla denatalità, che poi tanto semplice non è. Ma il fenomeno non è solo questo. Il fenomeno racchiude anche l'emigrazione giovanile. Parliamo di giovani dai diciannove una generazione che rappresenta il cuore di una Nazione; proprio quella fascia di età che incide notevolmente nell'economia di un Paese, stimolando anche l'indotto. Quindi, perché vederli fuggire e non iniziare, invece, a pensare insieme a una possibile soluzione? Come volevasi dimostrare, l'emendamento non è stato nemmeno tenuto inconsiderazione, ma vi è stata la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno. Non deve Non deve essere il contentino, però, l'ordine del giorno, per dare la possibilità a Tizio, Caio e Sempronio di fare un piccolo comunicato stampa per un momento di gloria. L'ordine del giorno, con la formula «a valutare l'opportunità di», è un investimento chiarissimo al Governo, che non può far finta di dimenticare o di conservare nel cassetto. Ciò significa che si spera che, nei prossimi provvedimenti, certe certe potenziali soluzioni possano essere prese in considerazione. E perché non pensare anche all'apporto che Fratelli d'Italia può dare in questa direzione? Sappiamo benissimo come Giorgia Meloni tutto il partito siano attenti a questa tematica, attenti alle necessità dei giovani e alle famiglie. Su questo mi ricollego a un'altra tematica, che abbiamo cercato di rappresentare con degli emendamenti risolutivi, ovvero quella dei docenti che chiedono da anni il rientro nei propri luoghi di provenienza. Si tratta di docenti che sono stati

l'anno scolastico è cominciato da tre mesi e, quindi, si sarebbe ancora in tempo. Voi vi chiederete che relazione c'è con l'inverno demografico: c'è, eccome! Noi abbiamo nuclei familiari divisi,

intersecate, giocano in armonia; per cui non permettere una vita serena ai docenti che hanno a che fare con delle risorse umane significherà chiaramente incidere anche negativamente sull'offerta formativa.

manifestare insensibilità nei confronti dei terremotati che attendono di rientrare nelle loro case.

è un'indennità di disoccupazione avente la funzione di fornire la tutela al sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (i dipendenti), vale in questa legge di bilancio, per il 2022, 250 milioni di euro. Pertanto, migliaia di lavoratori dipendenti del settore avranno la possibilità di usufruirne. Ricordiamoci sempre che nel settore agricolo vale il ricambio generazionale, perché molti giovani sostituiscono, anche e soprattutto per i lavori usuranti, i lavoratori dipendenti del settore agricolo. E questa è una funzione di accompagnamento e soprattutto soprattutto di aiuto e sostegno verso la pensione. Nel testo iniziale erano presenti misure molto importanti: la valorizzazione della competitività delle filiere,

poi l'emendamento sul reimpianto di piante resistenti alla *xylella*. È fondamentale dare ai territori interessati dei reimpianti alternativi importanti. al sostegno agli allevamenti degli animali da pelliccia (i visoni). Ringrazio il collega Bossi che si è molto impegnato in questo senso, come anche per il divieto delle emissioni di specie ittiche alloctone. Così facendo saremo in grado di ridare alla pesca nazionale un valore vero che si era perso nell'ultimo anno. Nessuno è stato in grado di metterci le mani: lo abbiamo fatto noi con questo emendamento che vale 150.000 euro per il 2022 e 150.000 euro per il 2023. Daremo le risposte ai nostri pescatori, grandi appassionati di territorio che sono anche i custodi dell'ambiente, perché in prossimità di dove pescano riescono anche a essere le sentinelle del territorio. Un altro emendamento importante,

ha avuto un problema enorme: da una parte, ha perso competitività a causa dei costi delle materie prime e dei costi energetici, anche e soprattutto negli allevamenti, nella logistica e nella trasformazione;

alla riduzione dell'accisa sulla birra; un valore importante, che permetterà ai nostri produttori di birra, autori di questo *made in Italy* straordinario, di produzioni vere, che tutti ci invidiano nel mondo,

Pensiamo anche all'emendamento che riguardava le quote latte: nel sistema del mondo allevatoriale questa è una piaga, perché le colpe dei padri ricadono sui figli. È un tema importantissimo che non dobbiamo sottovalutare,

Dall'altra parte, devo ricordare che noi abbiamo la forza, l'energia di fare le cose. Si poteva fare di più anche sulla fauna,

Mi sembrava che avesse concluso.

come tutti i provvedimenti importanti - ha avuto una gestazione faticosa e impegnativa, ma poi un'accelerazione perché - come dice l'antico motto - «alla fine il moto è più veloce», detto in italiano. Voglio sottolineare alcune misure, tra le tante, che riguardano il comparto sicurezza e difesa. Nel 2010 - c'era un Governo di centrodestra - fu sancita la specificità del comparto sicurezza e difesa; con quella legge di undici anni fa si volle stabilire il principio che gli appartenenti alle Forze dell'ordine non svolgono un lavoro come quello degli altri: è un lavoro molto più logorante, nel quale il rischio di perdere la vita è superiore rispetto a

senza risorse è un riconoscimento morale. Noi annunciammo che si sarebbero fatte delle scelte; ad esempio, il comparto fu escluso dall'applicazione della legge Fornero, perché non era ovviamente possibile applicare norme previdenziali con età di uscita troppo avanzata a chi svolge un'attività logorante. In questo disegno di legge voglio sottolineare l'articolo 27, che istituisce, proprio sul tema previdenziale, un fondo per interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco. Dobbiamo tutelare anche il loro destino previdenziale, perché comunque, con i calcoli che oggi si fanno delle pensioni, c'è il rischio che persone che hanno iniziato a lavorare ora vadano in pensione con assegni esigui. Sappiamo bene che gli stanziamenti economici non sono sufficienti, ma si è ma si è sancito un principio di specificità. L'articolo 27 va nel solco di quella legge del 2010, voluta dal centrodestra. Per la previdenza di queste persone, donne e uomini benemeriti, occorrono una perequazione, una integrazione, una possibilità di dar luogo a forme di indennità previdenziale integrativa. Ci sono degli stanziamenti per i prossimi anni, che dovranno essere integrati. Io mi auguro anche che venga approvata una proposta di legge che rafforzi questo indirizzo, che abbiamo sottoscritto insieme a tanti parlamentari di tutti i Gruppi; se n'è fatta promotrice la senatrice Pinotti e l'hanno firmato esponenti di tutti i Gruppi. Il provvedimento di cui all'articolo 27 va in questa direzione. Nel corso delle ultime ore si è molto discusso - ad esempio - sulle assunzioni per il comparto sicurezza e difesa e nella nottata ha preso corpo un emendamento che nasce da emendamenti che io stesso ho firmato, insieme ad altri colleghi di Forza Italia, ma che anche altri Gruppi hanno sostenuto e firmato. Si stanziano delle cifre significative per delle assunzioni che vadano a rivedere gli organici delle Forze di polizia. Ci sono stanziamenti che dal 2022 proseguono e si incrementano fino addirittura al 2032,

nazionali e alle Forze armate, che rientrano in queste misure e in tali provvedimenti. Nella legge di bilancio si interviene anche per rifinanziare alcune prestazioni dell'operazione "Strade sicure". I militari nelle strade non solo alleggeriscono le Forze di polizia di molti compiti, ma collaborano anche alle attività connesse all'emergenza del Cina virus. Il controllo del certificato sanitario richiede un maggiore impegno e una maggiore azione; giustamente i vertici del Viminale e di altri Ministeri avevano sollecitato degli interventi. La legge di bilancio dà delle risposte anche in questa direzione. Ed è quindi un fatto assolutamente positivo, al quale hanno contribuito molto l'azione di Forza Italia e quella unitaria di tanti settori del Parlamento. Ci sono quindi interventi sulla previdenza, in ossequio alla specificità, e interventi sulle assunzioni. Poi si è avviata un'iniziativa importante, con un altro emendamento approvato nelle ultime ore, frutto di emendamenti che il sottoscritto, Forza Italia e altri Gruppi hanno presentato, con una volontà molto ampia e trasversale: si è istituito un fondo per la tutela legale degli esponenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, attraverso polizze assicurative, per evitare che, a seguito di eventi dannosi (ma non dolosi ovviamente)

Noi riteniamo che nell'esercizio delle attività possano aprirsi delle controversie. Se c'è il dolo, ovviamente vale il principio penale, al quale nessuno è sottratto; ma in altri casi occorre che il personale che serve la sicurezza pubblica in divisa e può essere anche quello delle Forze armate, oltre a quello dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, possa essere tutelato e salvaguardato. È stato pertanto istituito questo fondo, con una tabella di ripartizione; c'è anche la Polizia penitenziaria in tutti questi provvedimenti e la voglio ricordare. Quindi c'è un intervento concreto; altro ancora si dovrà fare sulla tutela sanitaria e su altri capitoli. Vorrei sottolineare in questo intervento l'attenzione al comparto sicurezza e difesa, che del resto attende anche la conclusione del contratto. Con il nuovo Governo e con il ministro Brunetta si sono riaperte le trattative per il contratto, che scade alla fine di quest'anno.

scattiamo tutti quanti in piedi nei momenti di commozione e di omaggio all'impegno delle Forze di polizia o - Dio non voglia - quando accadono eventi tristi e drammatici. Noi diciamo sempre che non bisogna limitarsi agli applausi, ma bisogna passare ai fatti. In questo momento non c'è certo *pathos* emotivo, ma ci rigore operativo e concretezza nell'appostare delle risorse. Il nostro Gruppo, io stesso e altri colleghi, siamo sempre stati attenti a queste esigenze. il fattore sicurezza e il fattore popolo in divisa è uno degli elementi caratterizzanti. Ci sono però anche tanti altri aspetti. Voglio anche ricordare un'altra proposta che è venuta da Forza Italia - sicuramente ci saranno stati anche altri colleghi, ma io ricordo le nostre proposte emendative affinché la politica dei *bonus* per l'edilizia intervenisse anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche, aiutando il mondo della disabilità, di cui abbiamo parlato in queste ore approvando una legge delega con un coro di consensi doveroso,

nel tempo perché gli anni passano e a volte ereditare uno di questi immobili è più un guaio che un vantaggio. È infatti un onere fiscale ed è anche un dovere morale non abbandonarle. E allora nella politica dei *bonus*, che abbiamo fortemente sostenuto,

Oggi, grazie all'impegno di ciascuno di noi, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia e alla volontà di Giorgia Meloni, che ha deciso di dedicare tutta la dotazione finanziaria che aveva a disposizione per le libere professioni italiane, dopo venti anni di battaglie dopo venti anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria, delle casse di previdenza, i liberi professionisti hanno riconosciuto il diritto alla salute. Molti non lo sanno, ma purtroppo, fino a ieri, questo diritto non era riconosciuto ai liberi professionisti. I liberi professionisti che si ammalavano o si infortunavano dovevano non solo pagare le conseguenze dell'infortunio, ma addirittura pagare le conseguenze sanzionatorie dell'impossibilità di poter svolgere la loro professione. Dovevano quindi risarcire i clienti per le sanzioni che lo Stato comminava loro in conseguenza della malattia del professionista. Una cosa scandalosa, considerato che siamo in un epoca di civiltà; una cosa scandalosa che veniva da tutti additata e considerata come tale, ma che poi regolarmente non si riusciva a modificare.

una giornata per noi importante e un ringraziamento va a ciascuno di noi - mi sia permesso di dirlo - e ovviamente alla nostra *leader* Giorgia Meloni. voglio anche fare un ringraziamento cordiale, di cuore, sincero a ciascun parlamentare e soprattutto a ciascun membro della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, perché hanno dovuto rimanere ventiquattro ore, anche di più, bloccati in Commissione per cercare di arrivare di arrivare in Assemblea con degli emendamenti approvati e con un apporto del Parlamento a quello che il Governo aveva fatto.

nel quale i parlamentari, ossia le espressioni democratiche della vita politica, non avrebbero potuto dire una parola. parola. Ancora una volta, devo dunque dire grazie al mio partito e credo che sia tutto l'arco parlamentare a dover riconoscere all'opposizione costruttiva e seria di Fratelli d'Italia il fatto che abbiamo permesso alla maggioranza di arrivare in Parlamento con un lavoro svolto dalle Commissioni. Sarebbe bastato che un'opposizione, come tante ce ne sono state nel passato (mi basterebbe pensare alle opposizioni chiassose delle scorse legislature), avesse voluto fare del populismo e il Parlamento sarebbe stato completamente esautorato da ogni ruolo, lasciando al Governo l'assoluta e totale paternità della legge di bilancio: ricordo che è una cosa mai accaduta nella storia parlamentare.

senatore Pichetto Fratin, non ci siamo non per sua responsabilità - l'ho detto più volte ed è noto il rapporto di stima che ci lega - ma perché purtroppo non è accettabile che il Governo operi non pensando ai tempi necessari alla valutazione del Parlamento, non pensando al fatto che il Parlamento non ha solo il diritto, ma ha il dovere civico e politico di interagire con il Governo nella esecuzione, nell'approvazione, nel miglioramento delle leggi e, in particolare, di un provvedimento così fondamentale qual è la legge di bilancio. Non solo siamo in ritardo (il disegno di legge di bilancio è stato presentato il 12 novembre, veramente in ritardo), ma addirittura in questo mese non si è fatto nulla per far lavorare le Commissioni. Siamo arrivati a questa notte, al 20-21 dicembre, per vedere il primo voto della Commissione, ossia il primo voto del Parlamento sulla manovra di bilancio: una cosa inaccettabile. È inaccettabile per quei parlamentari che hanno dovuto fare degli orari assurdi, ma soprattutto perché, con tutta la buona volontà, non si può fare in una notte quello che si poteva fare in una o due settimane. inaccettabile finanche nei confronti degli impiegati e dirigenti dei Ministeri e degli organi dello Stato, che dovevano ovviamente dare il loro parere sulle proposte emendative e che sono stati costretti anche loro a lavorare male e e in fretta. Quanto al cosiddetto Governo dei migliori, spero tanto che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere e capire che gli organi parlamentari non sono un *optional* a disposizione di qualcuno, ma sono una necessità perché le istituzioni funzionino e svolgano il loro ruolo.

tempo e nel termine, con il Parlamento, non "a valutare l'opportunità di", ma a fare una certa cosa. Quella certa cosa, signor Presidente, era il rinvio della riscossione delle cartelle per rottamazione-*ter* e saldo e stralcio; un impegno che il Governo aveva preso con noi, quindi con gli italiani, per la legge di bilancio. Purtroppo,

quello che era stato sospeso per un anno e mezzo: è inaccettabile nel merito e nel metodo perché, quando prende impegni, un Governo li deve mantenere, Draghi o non Draghi; chiunque è obbligato a essere coerente con la parola data.

e ovviamente riconoscimento del valore della cessione del credito d'imposta? Vi chiedevamo solo questo, ve lo chiedevamo in tanti, e purtroppo avete fatto troppo poco anche in questa direzione. Il tempo non mi permette di dire altro; voglio comunque ribadire la nostra posizione su questi temi e richiamare il Governo prossimamente a un maggior rispetto delle istituzioni parlamentari.

Che sarebbe stata una manovra deludente c'erano tutti i presupposti, e, purtroppo, si verifica quello che avevamo anticipato:

teatrino veramente molto deplorevole, a nostro avviso, per un Parlamento che ha già una configurazione anomala, con una maggioranza del 95

di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza. Come hanno sottolineato tutti i colleghi che sono intervenuti, abbiamo cercato, come è nostro solito, di interpretare il ruolo di opposizione patriottica e di dare contributi qualificati. Dobbiamo dire, con orgoglio, che oltre al risultato che è stato rappresentato dal collega De Bertoldi, esprimiamo soddisfazione per il fatto che il Governo ci abbia finalmente finanziando anche la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Si tratta di un modello messo immediatamente in campo dal nostro governatore delle Marche, Acquaroli, che da mesi proponevamo al Governo, affinché fosse portato in tutte le scuole italiane.

ormai da troppo tempo aspettano risposta. C'è grande delusione per la parziale proroga

risposta ai direttori generali dei servizi amministrativi, con un aumento della loro indennità amministrativa.

essere immessi in ruolo e a riempire gli spazi disponibili - che ci sono - per fare in modo che la scuola italiana abbia personale adeguato, visto soprattutto quanto ha subito negli ultimi tempi.

modo sono molto deludenti gli interventi che riguardano la cultura e lo sport, di cui ha già parlato il collega Barbaro.

assistere ad un'elezione in cui i politici votano altri politici, nell'indifferenza dei cittadini, è veramente mortificante, quando questi enti hanno ancora funzioni fondamentali, che riguardano le scuole e le strade provinciali. Il piano da 510 milioni di euro, per 94 enti, spalmato in tre anni, non rappresenta dunque assolutamente una risposta risolutiva.

con cui a nostro avviso si paga una cambiale elettorale, che però non salva né Napoli, né altre città, perché è evidente che per fronteggiare il gravame che viene da anni di squilibri amministrativi occorrerebbero ben altri interventi, per fare in modo che queste realtà amministrative, che rappresentano

un giudizio estremamente negativo sulla manovra. Come ha detto la senatrice Rauti, un'operazione di ragioneria, ma aggiungerei anche, in alcuni casi, di salumeria, viste le mancette che sono previste all'interno del testo. A prescindere da chi sarà il nuovo Capo dello Stato, è evidente che questo Governo, con la sua contrastante maggioranza, ha esaurito la sua vita e sembra sempre di più un gigante dai piedi d'argilla.

trepidante attesa. Devo dire che la condizione è eccezionale, anche perché il Governo è rappresentato autorevolmente

che entra in un momento particolare della vita degli italiani. Prima uno dei relatori, il senatore Vasco Errani, ha definito questo un momento di crescita inaspettata. Probabilmente era una crescita da programmare, o meglio, una crescita che qualcuno aveva pensato di programmare.

è stato uno strumento che ha portato via decine di migliaia di persone da questa terra, ha sacrificato famiglie, ha sacrificato in un momento storico un'economia già ammalata, ma ha aperto ma ha aperto gli occhi ad un sistema politico, nazionale, europeo ed internazionale, sul fatto che probabilmente i sistemi economici pensati, controllati e regolamentati fino a quel momento, non avevano più ragione di esistere. Aver sbloccato un sistema, purtroppo soltanto dopo una grave problematica quale la pandemia, ha causato un rimbalzo economico

noi dobbiamo essere capaci di coglierlo e renderlo strutturale. Ora, pensare che l'Italia possa crescere nei prossimi cinque anni del 6,2 per cento significherebbe avvicinarsi alla crescita degli ultimi dieci anni della Repubblica Popolare Cinese, il che mi parrebbe quantomeno un po' difficile e complicato. Tuttavia, le misure messe in atto e i sistemi che sono stati smontati e che hanno consentito una valorizzazione del sistema economico nazionale ed europeo, devono servire alla strutturazione delle imprese, della nostra società e a renderci seriamente interessati al futuro, non al presente. Cito nuovamente il collega Errani nel suo intervento introduttivo, quando ha detto

per un futuro consolidato di un'economia che ovviamente ha un'opportunità. Allora, dobbiamo essere noi imprenditori - mi ci metto anch'io, seppur piccolissimo - a guardare avanti con senso di responsabilità. Abbiamo lavorato molto bene. I *bonus* di cui parlavo poco fa valgono nell'edilizia complessivamente probabilmente oltre 100 miliardi di euro. Sono stati mantenuti liberi da vincoli e vincoletti; è stato fatto molto per evitare delle crisi che si sarebbero verificate. Abbiamo dato una spinta al turismo e alla cultura;

abbiamo un'opportunità; abbiamo lavorato bene insieme, seppur con difficoltà e con opinioni diverse; cerchiamo di fare in modo che il Paese capisca e che noi capiamo che questa è un'occasione che non possiamo perdere.

Governo, colleghi, la discussione odierna verte sulla legge più importante che ogni anno il Parlamento si trova ad approvare, la legge di bilancio. Il provvedimento già in partenza era buono, ma che, come ogni volta, sarebbe stato possibile migliorare e per questo avevo presentato oltre 30 emendamenti a mia firma.

presente nel nostro sistema per cui i *pickup*, essendo immatricolabili solo come autocarri, possono essere utilizzati solo per l'esercizio dell'attività di impresa e, quindi, potrebbero trasportare solo gli addetti legati all'attività di quell'impresa. Noi, invece, sappiamo benissimo che vengono abitualmente utilizzati per il trasporto di persone, con il rischio che, nel caso di incidente, i trasportati non sarebbero coperti. Chiedevo di eliminare questa anomalia. Sarebbe costato zero allo Stato e quasi sicuramente ci sarebbe stato un gettito per l'erario, un introito perché, non essendo immatricolabili per scelta - l'attuale possibilità sarebbe rimasta come autocarri, non ci sarebbe stato il recupero dell'IVA, né la detrazione delle spese sostenute. Sarebbe stato addirittura un vantaggio fiscale per lo Stato e avrebbe eliminato un problema che purtroppo riguarda centinaia di migliaia di mezzi. Vista la mia provenienza, come era lecito e logico aspettarsi, la maggior parte degli emendamenti riguardava il terremoto. Peccato che non sia stato approvato il provvedimento con cui si chiedeva la deroga per il calcolo delle piante organiche delle scuole del cratere. Era un provvedimento che avevo ottenuto da sindaco già nell'ottobre 2016, quando in occasione di un incontro con l'allora presidente del Consiglio Renzi ad Arquata del Tronto evidenziai che molte delle persone costrette ad andarsene dai nostri luoghi avevano dei figli che inevitabilmente avrebbero iscritto in altre scuole e che, quindi, serviva una deroga per evitare che la riduzione dei servizi offerti portasse quelle persone a non rientrare più. Purtroppo è un problema che non è stato risolto. è un peccato non aver accolto un emendamento a prima firma del collega Briziarelli con cui si chiedeva l'istituzione di un osservatorio sui terremoti e su come era stata poi gestita la ricostruzione. Già tre anni fa, in Commissione, avevo chiesto di avviare l'*iter* per una legge di gestione delle emergenze. Questo perché, avendone vissute diverse direttamente sulla mia pelle, so perfettamente, anche da *ex* amministratore locale, quanto sia difficile, inopportuno e sconveniente dover ricominciare ogni volta daccapo, senza nemmeno sapere quali sono i ruoli. Quindi, approvare una legge di gestione delle emergenze prima, in tempo di pace, sicuramente ci consentirebbe di farci trovare pronti quando, purtroppo, si verificherà un'altra emergenza. Invece, la legislatura sta per finire, a prescindere se la sua scadenza sarà naturale o anticipata, e temo proprio che arriveremo alla fine della legislatura senza che questa legge sia approvata. Peccato. È per me un rammarico importante - infatti ogni volta presento questo emendamento - che non sia stato risolto il problema costituito dall'articolo 10 del decreto n. 189 del 2016, poi convertito nella legge n. 2016, che comporta l'assurdo per cui la ricostruzione di alcuni privati sarà pagata da altri privati. La proroga del superbonus sospende e rinvia questo problema, spostandolo alla fine del 2025 ma non risolvendolo. Quindi, prima o poi prima o poi andrà risolto. Così, però, ho già introdotto una delle misure che, invece, mi soddisfano molto, appunto la proroga del superbonus per le aree terremotate. Da subito avevo evidenziato la necessità di questa proroga. Innanzitutto per motivi di equità, perché per me era assurdo creare la sperequazione per cui chi sceglieva discrezionalmente di fare un intervento usufruendo dei *bonus* non pagava nulla, mentre chi, invece, era costretto a fare l'intervento per causa di una calamità naturale si ritrovava ad avere degli accolli. equità, dunque, era giusto e opportuno che questo *bonus* venisse prorogato, anche perché nei comuni terremotati spesso ci si trovava nell'impossibilità di poter presentare i progetti. Pensiamo alle aree perimetrate perché all'interno dei centri storici distrutti; pensiamo alle aree interessate da un PSR, un piano speciale di ricostruzione. Tutte condizioni oggettive, impedimenti oggettivi, anche solo per la presentazione del progetto, quindi figuriamoci per rendicontare entro i termini previsti dalla legge. Era dunque necessario che questi *bonus* venissero prorogati, anche a causa dell'aumento enorme del costo delle materie prime, che ben conosciamo, perché ha già inciso direttamente sulle tasche di tutte le famiglie italiane e, purtroppo, ancora lo farà nel futuro. Tale aumento ipotizzati inizialmente purtroppo non siano più attuali. Quindi, è una necessità oggettiva per la ricostruzione. Ovviamente ci sono altre soluzioni, chieste e ottenute, come ad esempio segnali di attenzione per i Comuni, come ad esempio segnali di attenzione per le attività produttive, che si ritrovavano nella condizione di dover anticipare per intero il costo dell'IVA. Tutte soluzioni che erano necessarie e che hanno avuto accoglimento in questa manovra. Approfitto del tempo che rimane manovra. Approfitto del tempo che rimane per uno spunto di riflessione che propongo a tutta l'Assemblea. La ricostruzione non deve rimanere fine a se stessa. Purtroppo, in quelle aree abbiamo perso una generazione, perché molte persone, quasi tutte, sono state costrette ad andarsene nell'imminenza del terremoto. Molti di coloro che avevano dei figli, li hanno iscritti a nuove scuole, da cui poi non avrebbero potuto sradicarli per rientrare nei Comuni di appartenenza; altri sono stati costretti a trovare lavoro fuori; ad andarsene per i motivi più disparati. Comunque, noi abbiamo perso delle persone e questa generazione persa, in Comuni che hanno già decremento demografico, rischia di diventare mortale.

L'innovazione, da sempre al centro dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle, e l'originalità contraddistingueranno sempre più le scelte di politica economica del MoVimento 5 Stelle. L'innovazione, come si sa, spiazza un po' tutti: all'inizio non è possibile comprendere il pieno potenziale di una misura, in che modo sarà capace di contribuire.

si chiedevano come era possibile che si potessero realizzare interventi a costo zero perseguendo l'obiettivo ambientale del risparmio energetico. Certo,

Non abbiamo certo pensato che potesse essere facile, nella misura in cui poche persone avevano sin dall'inizio capito quel meccanismo virtuoso, quella innovazione introdotta con il superbonus 110 che dobbiamo tutti ricordare. Mi riferisco al meccanismo dello sconto in fattura e della certificazione, cessione e circolazione del credito a tutti gli altri *bonus* edilizi. Questo è il vero valore, questa è la vera chiave di lettura del superbonus 110

che in termini di investimenti dovuti al superbonus significano 12 miliardi di euro (più 6.200 per cento rispetto all'inizio dell'anno). Secondo l'ultimo rapporto sull'impatto degli incentivi fiscali in edilizia, elaborato dal Servizio studi della Camera con il Centro tra superbonus e vari altri *bonus* edilizi sono stati generati lavori incentivati per 51 miliardi di euro (più 82 per cento rispetto al 2020). Questo significa in primo luogo che sono stati creati 510.000 posti di lavoro in secondo luogo che ci siamo avvicinati molto agli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima in termini di risparmio energetico. Un ultimo studio fatto dal Consiglio nazionale degli ingegneri afferma che il superbonus

Infine, uno studio di Unioncamere-Infocamere afferma che negli ultimi due anni sono state costituite ben 30.000 nuove imprese di costruzioni. Potrei ancora procedere con i dati, ma preferisco fermarmi e capire dove stiamo andando. Che questa sia la direzione giusta ce lo ha certificato la stessa Commissione europea con alcuni suoi rappresentanti, come il vice presidente Timmermans e la commissaria Simson,

possiamo però passare ai contenuti del disegno di legge di bilancio che, assieme al decreto-legge antifrode, hanno finito per disorientare alcuni operatori. Purtroppo alcune misure hanno finito per discriminare alcuni interventi rispetto ad altri, come pure si poteva temere ingessassero il meccanismo. Il MoVimento 5 Stelle ha proposto un pacchetto di emendamenti (parliamo di oltre 20 emendamenti soltanto sul superbonus) che ha condiviso con le altre forze di maggioranza ed è riuscito a formulare una serie di proposte che il Governo ha in larga parte accettato. Finalmente potremo contare sui seguenti risultati. Il primo, tanto atteso, è la proroga al 2022 del superbonus sulle case unifamiliari, senza alcun riferimento al tetto ISEE, alla CILA e all'abitazione principale, purché

nelle aree colpite da sisma *post* 2009. Il terzo è l'allineamento della scadenza dei lavori trainati come per quelli trainanti, importante per migliorare di due classi energetiche l'efficientamento energetico della casa, come pure riconoscere le spese delle asseverazioni all'interno delle detrazioni fiscali previste dai *bonus.* abbiamo così restituito al superbonus l'ampiezza che meritava. In questo modo sarà in grado di continuare a sprigionare tutta la sua potenzialità in termini di crescita economica, generazione di posti di lavoro e tutela dell'ambiente.

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (2483). Il provvedimento è stato assegnato alla 5ª Commissione,

confermato fino alla fine. Veramente non serviva scomodare Draghi per una tale legge di bilancio. Ci sono un problema nel merito e uno nel metodo. Il disegno di legge di bilancio

la notte più lunga dell'anno e anche molto buia per il Senato, vedendo come è ridotto.

I giornali già ne hanno pubblicate diverse, visto che ce ne sono di svariate e vergognose: 82.000 euro per l'assunzione di due dipendenti in un piccolo Comune e un milione di euro per la ristrutturazione della palestra di uno specifico Comune. Un milione di euro per l'efficientamento energetico della piscina comunale di un Comune, che sarà di un senatore della maggioranza. Veramente da vergognarsi, e non solo per questo,

Fratelli d'Italia a questo squallore, però, non è sceso. Abbiamo battagliato, soprattutto grazie ai nostri senatori in Commissione bilancio, per tentare di migliorare il testo. Con le nostre poche forze disponibili al Senato qualcosa abbiamo fatto; i miei colleghi lo hanno già raccontato e lo racconteranno anche domani. Penso al diritto finalmente esteso ai liberi professionisti di ammalarsi, senza che questo comporti la la mancanza degli adempimenti tributari ai quali sono tenuti; penso alle risorse destinate alla ventilazione meccanica per l'areazione delle scuole. Il Covid-19, infatti, soprattutto dove non c'è ricircolo d'aria: nelle scuole serve la ventilazione meccanizzata, non servono altre sciocchezze. *(Applausi)*. Lo abbiamo detto e ripetuto e siamo riusciti a stornare parte dei fondi inutilizzati destinati alle scuole per realizzare

tutte le tasse su quell'immobile: la quota Irpef, la quota IMU, se non è prima casa, e la quota Tari. Grazie a Fratelli d'Italia, da quando viene fatta la denuncia di occupazione dell'immobile a quando quell'immobile non viene liberato, le le tasse sull'immobile occupato non saranno dovute. Questa era la battaglia che poteva e doveva fare il Parlamento in Commissione e non il riscaldamento della piscina del Comune di uno dei senatori.

Abbiamo proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come abbiamo il superbonus per gli ammortamenti, facciamo il superbonus per chi assume persone in Italia. Questo agevola l'economia reale e sfavorisce le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere: bocciato l'emendamento. Purtroppo Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del Covid-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti,

ponendo a carico dello Stato il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. È un meccanismo che, per esempio, già funziona per l'occupazione femminile o l'occupazione giovanile. Anche questa ci sembrava una misura semplice, immediata e di buon senso,

posso tranquillamente non versare un euro allo Stato prima di ventiquattro mesi, non facendo qualcosa di illegale, ma semplicemente applicando la legge. Però, se io alla fine dei due anni sparisco, il fisco non mi rintraccia più. ci sono delle piccole accortezze che si possono adottare: per i soggetti a rischio, prevalentemente chi è extracomunitario (non perché uno voglia fare discriminazione, ma perché è più facilmente non più reperibile), fare un fondo un fondo cauzionale o una fideiussione sulle tasse che saranno dovute. Un'altra cosa a costo zero per chiunque è l'obbligo di PEC per gli amministratori di società. Noi abbiamo un sistema nel quale c'è l'obbligo di PEC per le società, ma non c'è l'obbligo di PEC per gli amministratori delle società. Questo vuol dire che prendo una testa di legno, gli faccio fare la società, dopo i due anni chiudo, sparisce la società, non ho pagato un euro e non c'è neanche la possibilità di notificare l'atto. Non notificare l'atto vuol dire che, per esempio, il dipendente non pagato non ha neanche diritto a rifarsi all'INPS per il TFR non pagato. Perché ci avete bocciato la richiesta di obbligo di PEC per gli amministratori di società? Costava zero, avrebbe aiutato a combattere la concorrenza sleale e avrebbe aiutato i lavoratori. Purtroppo il tempo è finito e gli argomenti erano molti. solamente che Fratelli d'Italia pensa che all'Italia servano crescita e lavoro; per fare questo va aiutato il nostro tessuto produttivo. di legge di bilancio non lo fa ed è purtroppo un'occasione persa, non per Fratelli d'Italia, ma per la Nazione.

in Parlamento di questa manovra. L'*iter* di questo disegno di legge è apparso già segnato ben prima di cominciare. È sicuramente una legge di bilancio che prenderà qui la la fiducia e arriverà blindata alla Camera. Per quanto riguarda la questione di merito, una delle cose importanti

esistenti, e neanche ai contribuenti, che sono perseguitati dall'Agenzia delle entrate. C'è stato un taglio delle tasse di 8 miliardi, che sarà poco incisivo, mentre sarà finanziato il reddito di cittadinanza. È un documento che non ha nessun tipo di

la burocrazia ha limitato molto le risposte. Nell'ultimo anno e mezzo sicuramente c'è stata una volontà da parte delle piccole e medie imprese, che hanno avuto nel superbonus cento solamente la possibilità di vedere incrementata la loro redditività; purtroppo il Governo non è riuscito a dare delle risposte importanti. Anche per quanto riguarda il merito della questione relativa allo stanziamento di risorse, occorre sottolineare che si continuano a finanziare - come dicevo prima - delle spese improduttive per il Paese, come il reddito di cittadinanza (anche se forse è stato un po'

nella formulazione attuale prevista in questo disegno di legge di bilancio prevede soprattutto delle forti limitazioni. *In primis,* la proroga

subisce un calo con il passare degli anni, chiaramente questa misura non è sicuramente attrattiva. Sempre per quanto riguarda il tema del superbonus, ho presentato personalmente, insieme

che sicuramente la maggioranza non ha avuto coraggio e non ha avuto una visione per il Paese soprattutto perché ci sono state queste liti che hanno ritardato molto l'approvazione del bilancio. Un documento che senza avere nessun tipo di visione politica sicuramente creerà dei problemi nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni. Noi come Fratelli d'Italia saremo vigili per migliorare, ove possibile, tutti i provvedimenti, in questo caso presentando degli emendamenti che possano migliorare

il Presidente della Repubblica la settimana scorsa ha consegnato gli attestati d'onore di alfiere della Repubblica, conferiti a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza che si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento. È con grande piacere e forte commozione che porto all'attenzione del Senato e della Nazione la nomina ad alfiere della Repubblica di Antonio Maria Granieri, premiato con la motivazione di essere diventato testimone di socialità e amicizia nell'attività dell'associazione «Down Dadi» di Padova, nel sostegno ai compagni che hanno bisogno di maggiore aiuto nel dialogo con i coetanei. Antonio è un ragazzo di diciotto anni di Vigonza, in provincia di Padova; è solare e socievole. La sua famiglia è composta da mamma Angela, papà Francesco, la sorella Teresa e la gemella Maria Elisabetta. Poi nonni, zii e cugini, lo avvolgono con tutto il loro amore. Frequenta il quarto anno dell'Istituto alberghiero di Abano, gli piace andare a scuola perché così può stare con i suoi compagni e divertirsi con loro, soprattutto durante il laboratorio di cucina. Nel tempo libero pratica due sport, ballo e baskin (basket inclusivo). Quasi ogni settimana frequenta «Casa Vela», un progetto di autonomia dell'Associazione «Down Dadi» di Padova. È qui che ha incontrato i suoi migliori amici. Un suo difetto è la testardaggine, ma questo lo porta a voler sempre trovare un modo per aiutare i suoi amici in difficoltà. I suoi pregi più belli sono infatti la bontà e l'altruismo verso chiunque, coetanei e non. Un piccolo dettaglio: Antonio ha la sindrome di Down. Nella società dello scarto sarebbe relegato ai margini, invece è la dimostrazione vivente che amati, stimolati e valorizzati dalla famiglia e da chi ci sta vicino, tutti possiamo essere felici e preziosi per la comunità. comunità. Antonio è icona dell'uomo che nella difficoltà sa valorizzare il disagio e si fa prossimo a chi soffre o non ce la fa. Parafrasando don Tonino Bello, Antonio è un ragazzo con una sola ala che abbraccia il fratello, anch'esso con una sola ala, e assieme si librano verso le vette più alte, quelle che rendono la vita degna di essere vissuta.